recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Si tratta di una tematica di scottante attualità e di grande valenza, che rappresenta una questione cruciale per il futuro tecnologico ed economico della nostra Nazione, con significative refluenze, anche dal punto di vista geopolitico, che non sfuggiranno a nessuno. Questi materiali, infatti, sono essenziali per la produzione di tecnologie avanzate nei settori della difesa, aerospaziale e della transizione energetica. la domanda è destinata ad aumentare in maniera assolutamente esponenziale, ma l'Europa e l'Italia sono quasi totalmente dipendenti dalle importazioni e ciò le rende vulnerabili a significativi rischi di approvvigionamento. Basti pensare che il 97 per cento del magnesio utilizzato in Europa viene acquistato dalla Cina e il 63 per cento del cobalto mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, il 60 per cento del quale è raffinato in Cina. È questo il motivo per cui si sente forte l'esigenza di garantire all'Unione europea e all'Italia un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, data l'importanza per il funzionamento del mercato interno di questi prodotti, snellendo e sburocratizzando i termini e le procedure per il rilascio di titoli per l'estrazione e, al tempo stesso, per l'autorizzazione di progetti per il riciclaggio di materie prime. Veniamo all'esame dettagliato del decreto-legge in conversione. L'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo di definire, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1252, introducendo disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche. In questo ambito, ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ragione del preminente interesse nazionale all'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal più volte citato regolamento, sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche di cui all'articolo 2. Si ricorda che il 4 ottobre 2023 la 9ª Commissione ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento relativo alle materie prime critiche. L'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione e riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche. Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione e i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali. La concessione comporta, ove richiesto al concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica. Per i progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche. Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche e i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione da parte del punto unico di contatto. L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quale la Conferenza dei servizi. L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia. L'articolo 7 al comma 1 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) a valutazione di incidenza, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma. Il permesso di ricerca dev'essere comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'articolo 8 impone, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici, il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto fra il 5 e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati a essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione interessata per i progetti su terra ferma. L'articolo 9 è volto a incrementare il recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. L'articolo 10 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il compito di elaborare il programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si dispone che la carta mineraria, aggiornata sulla base delle risultanze del programma nazionale di esplorazione, venga pubblicata sul sito dell'ISPRA entro il 24 maggio 2025. L'articolo 11 stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*. A tali fini, si istituisce presso il medesimo Ministero il registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. L'articolo 13 reca norme volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. L'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Mimit

già richiamati dalla norma originaria, operando, ai fini della loro individuazione, un richiamo ai relativi codici della nomenclatura tariffaria europea. L'articolo 14-*bis* detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy non ricomprese nel citato Regolamento

modifica l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, prorogando dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo pari a 2,525 miliardi

desidero fare, a nome di questa Presidenza, gli auguri di buon compleanno alla senatrice Tubetti e al senatore Enrico Borghi.

il decreto-legge n. 84 del 2024, oggi all'esame dell'Assemblea, rappresenta una trasposizione, sia pur non completa nella realtà nazionale, del Regolamento (UE) 2024/1252 sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche per l'industria europea. Il suo obiettivo è quindi quello di disciplinare le procedure, attribuire le competenze e definire i meccanismi per garantire una fornitura di materie prime essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica veicolare e soprattutto digitale. Uno degli attori principali dell'attuazione di quanto previsto dal decreto è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca che è quello di ricostruire le basi conoscitive per la definizione del potenziale minerario nazionale tramite la redazione e realizzazione dell'importante programma nazionale di esplorazione generale, richiesto dall'articolo 19 del regolamento europeo, compito reso complicato dal progressivo abbandono, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, per motivazioni di carattere economico, ambientale e sociale, delle attività minerarie di minerali metalliferi, cioè dei materiali che oggi sono indispensabili per il nuovo modello di sviluppo decarbonizzato.

che rappresenta il punto di partenza per i compiti affidati all'Istituto dal decreto-legge n. 84. Nel *database* sono infatti contenute le informazioni basate sui dati pregressi relative alle risorse minerarie nazionali. In passato sono stati coltivati diversi giacimenti di quelle che oggi sono considerate le materie prime critiche. Attualmente però solo in 22 miniere, delle 76 attive, si estraggono materie prime critiche; in venti di queste si estrae il feldspato, minerale essenziale per l'industria della ceramica, e in due la fluorite, che ha un largo consumo nell'industria dell'acciaio, dell'alluminio, del vetro, dell'elettronica e della refrigerazione. Per quanto riguarda i metalli, il nostro Paese risulta ad oggi totalmente dipendente dai mercati esteri, ma esistono ancora delle potenzialità per la mitigazione di tale dipendenza. Esiste infatti nel territorio italiano la potenziale la potenziale presenza di materie prime critiche e strategiche come il litio, scoperto in quantitativi importanti nei fluidi geotermici tosco-laziali e campani, e diversi altri minerali da cui si producono metalli indispensabili per il modello di sviluppo decarbonizzato, la *green tech*, la transizione digitale. Depositi di rame, manganese, tungsteno, cobalto, magnesite, bauxite, barite, fluorite e terre rare potrebbero essere rivalutati grazie alle nuove tecniche di esplorazione e di gestione sostenibile delle attività minerarie, supportate dall'andamento favorevole dei prezzi di mercato. In questo contesto si inserisce il programma nazionale di esplorazione generale, che l'Italia ha l'obbligo di realizzare e che ha lo scopo di identificare le aree minerarie più promettenti e di fornire elementi di base utili a incentivare l'interesse da parte delle compagnie minerarie a richiedere i permessi per svolgere una ricerca mineraria operativa e completa. È proprio sull'articolo 10 del decreto-legge in esame che vorrei soffermarmi, in particolare sulla tempistica di attuazione del programma nazionale di esplorazione.

mentre, in realtà, l'articolo 19 del regolamento non pone un termine definito alla completa implementazione delle misure pianificate del programma, anche se si può presumere che debbano essere concluse al momento della prevista revisione del programma, cioè dopo cinque anni. Certamente bisogna adempiere all'informativa sullo stato di attuazione nell'ambito del *report* annuale, quindi la data di presentazione anticipata al 25 marzo 2025 2025 è molto impegnativa per noi. Tale testo lascia intendere che in due mesi l'ISPRA dovrebbe fare un lavoro per il quale servono tempi più lunghi e condizionati anche da un apparato burocratico

l'esecuzione delle campagne di ricerca e la restituzione dei risultati delle analisi siano assolutamente impossibili per il 25 maggio 2025, cioè dopo due mesi dalla presentazione del programma. Si chiede di far sì che venga prodotta questa cartografia definitiva basata sui risultati delle ricerche, che notoriamente hanno tempi più lunghi. Occorrerebbe pertanto in un prossimo provvedimento rivedere questo passaggio, scrivendo che la carta mineraria dovrà essere sottoposta ad aggiornamenti annuali sulla base dell'avanzamento delle ricerche. L'articolo 19 del citato regolamento prevede, tra le azioni da intraprendere per realizzare il programma nazionale di esplorazione, anche la rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti. Tale punto è stato inserito al comma 8 dell'articolo 10, cui l'ISPRA ha ottemperato il 24 luglio 2024, aprendo al pubblico il *database* minerario nazionale: un'azione molto importante. Tale attività non può però essere considerata conclusa, ma è in continua evoluzione con il procedere dell'attività di recupero delle informazioni pregresse. Il tema del comma 9 dell'articolo 10 riguarda anche l'aspetto finanziario. Infatti, nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, se ne stima uno medio per singola area di circa 150.000 euro. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi, la cui necessità sarà valutata caso per caso. caso. Appare evidente che, con il finanziamento importante che è stato messo in campo dal Governo, pari a 3,5 milioni di euro, al netto delle altre spese per la realizzazione del progetto, gli studi previsti dal programma nazionale potranno essere eseguiti su non più di venti aree del territorio nazionale, con l'estensione ognuna dell'ordine di qualche decina di chilometri quadrati. Conseguentemente, non potranno essere eseguite nuove campagne esplorative, per esempio sui fondali marini, come previsto dall'articolo 3, comma 8, a meno dell'esecuzione di eventuali analisi tramite altri progetti *in itinere*. Con queste cifre in gioco, è evidente che il numero di quaranta aree che ancora compare sul *dossier* iniziale, che ho letto con attenzione, è da considerarsi un auspicio più che una certezza. Sulla base di un presunto finanziamento, ci vorrebbe quasi il doppio di quanto realmente concesso dal decreto-legge in esame. Il mio auspicio, infatti, è che nella legge di bilancio ci metteremo mano, ma faccio appello all'attenta sottosegretaria Bergamotto, perché ha anche questa capacità di trasferire le informazioni di quest'Assemblea al Governo. Io credo, infatti, che questa sia un'attività molto importante e molto attesa. Vorrei sottolineare anche un miglioramento significativo dell'impianto apportato alla Camera dei deputati, che consiste nell'introduzione degli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattiva nelle attività di vigilanza e controllo sui permessi di ricerca per materie prime critiche, insieme all'ISPRA e alle sovraintendenze territorialmente competenti. Tra l'ISPRA e le Regioni non c'è questo divario questo divario di vedute: hanno tradizionalmente un forte legame, sia tramite il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, sia tramite la rete italiana dei servizi geologici. Vorrei poi fare un esplicito riferimento anche alla questione relativa all'estrazione mineraria dai fondali marini, ritenendo utile allineare il decreto alla posizione di grande cautela tenuta dall'Italia tramite il MAECI, di indirizzare prima di tutto l'attività alla ricerca mineraria. L'obiettivo che si è dato il Governo, emanando questo decreto-legge è stato quello, condiviso da questa maggioranza, di individuare le misure urgenti per la definizione di un sistema di gestione delle materie prime critiche che sono considerate strategiche. L'importanza è data dai numeri. Ci sono settantasei miniere ancora attive nel nostro Paese tutti i materiali che potremmo estrarre sono almeno diciassette: noi oggi ne estraiamo solo due. Per tutte le altre materie prime critiche necessarie per la transizione energetica industriale dipendiamo, come ho detto in precedenza, dall'estero. La mancanza di accesso diretto a queste materie prime può rendere le nostre aziende meno competitive, come sappiamo bene. Perciò andiamo avanti, signor Presidente, per ridurre questa dipendenza, dare forza all'estrazione interna, salvare l'utilizzo delle nostre risorse e concentrarci su una politica industriale seria e concreta, come seria e concreta è l'azione di questo Governo. *(Applausi)*. sia importante l'approvvigionamento delle materie prime critiche e di interesse strategico, in particolare per il futuro, in funzione della transizione energetica e anche climatica, se vogliamo considerarlo da questo punto di vista. Purtroppo, però, stati accolti alcuni emendamenti che noi abbiamo presentato alla Camera, questo decreto-legge non affronta una serie di questioni: anzi, ne ha affrontate alcune, espropriando il potere ad altri, in particolare, ovviamente, nel merito e nel metodo.

la questione della partecipazione, quando si affrontano problemi quali l'estrazione dal territorio di un prodotto, nel senso che le competenze vengono calpestate. Mettetevi d'accordo: siete per l'autonomia differenziata, ma, in questo caso, avete deciso di centralizzare tutto, calpestando ovviamente il ruolo delle Regioni. Vorrei però che tra di noi discutessimo anche di quello che avviene oggi. Già oggi, il fatto stesso che le Regioni abbiano il compito di decidere dove e in che modo estrarre, escludendo il ruolo dei Comuni e delle comunità locali, un problema grossissimo. Lo sapete tutti: chi fa l'amministratore sa che, molto spesso, i comitati vanno dal sindaco e la ricaduta l'hanno i Comuni

La montagna è squarciata, i lavoratori sono a casa e chi si è visto si è visto. Chi paga questo prezzo? Lo paga tutta la collettività, il territorio e tutti noi.

Governo, inizio il mio intervento descrivendo in maniera sintetica il contesto nel quale il provvedimento in discussione andrà ad operare. A livello europeo, esiste una serie di materie prime non agricole e non energetiche che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione della transizione verde e della transizione digitale, legate alle energie rinnovabili e all'industria digitale, con un ruolo importante nell'industria aerospaziale e della difesa. Ebbene, queste sono considerate materie critiche, in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi, con una domanda destinata ad aumentare in misura esponenziale. Se poi consideriamo le crescenti tensioni geopolitiche e gli scenari bellici che ci circondano, il rischio di difficoltà del relativo rifornimento necessariamente aumenterà in misura preoccupante. Non è finita qui, perché dobbiamo considerare anche i cambiamenti climatici, caratterizzati sempre più da eventi meteorologici estremi: c'è l'innalzamento del livello del mare, c'è la perdita delle biodiversità. ragioni, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali molto negativi. In questo contesto, l'Unione europea, attraverso il Regolamento n. 1252 del 2024, ha espressamente evidenziato che le azioni individuali dei singoli Stati membri, se non coordinate, non sono sufficienti a prevenire efficacemente le difficoltà di approvvigionamento di queste materie, per di più se vi è una regolamentazione inadeguata rispetto agli operatori di mercato. Per scongiurare questi rischi, il regolamento europeo ha espressamente indicato la necessità di diversificare il rifornimento di queste materie, rafforzando quindi la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri, al fine di garantire una sana competitività

come punto unico di contatto nazionale la direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provocando così un capovolgimento dell'assetto attuale delle competenze tra Stato e Regioni. Analoga centralizzazione riguarda poi il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici, con l'individuazione quale punto unico di contatto nazionale dell'unità di missione questa volta presso il Mimit. Il testo, poi, contiene anche norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie, disponendo che, per l'attribuzione della qualifica di progetto di interesse pubblico nazionale, nella stessa logica di concentrazione di poteri in capo al Governo, la competenza dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti sia istituita sempre presso il Mimit. Il decreto-legge poi istituisce sempre presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico permanente, un organismo molto importante, al quale sono affidate funzioni altrettanto importanti: si parla del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento; dovrà predisporre ogni tre anni un piano nazionale delle materie prime critiche, misurare il fabbisogno nazionale e istituire il Registro nazionale delle aziende e delle catene di valore strategico. Noi, però, ci chiediamo come si fa a definire necessaria e urgente l'individuazione di una disciplina di tipo ordinamentale, che prevede addirittura la costituzione di organismi così importanti. Questa potrebbe sembrare l'anomalia più importante, e invece no. La grave pecca che riscontriamo in questo decreto è il vero e proprio allontanamento delle Regioni interessate, di fatto scavalcate, completamente snobbate. Presidente, un decreto legislativo anziché un decreto-legge avrebbe garantito un adeguato coinvolgimento delle Regioni in seno alla Conferenza unificata per l'espressione quantomeno di un'intesa, e invece no. Ritorno sull'ennesimo abuso dello strumento della decretazione d'urgenza, con un Parlamento sempre più esautorato dei propri poteri, le minoranze vestite di un mero ruolo di testimonianza, nonostante le proposte opportune che abbiamo presentato. Per ciò che riguarda il merito, consideriamo sicuramente indispensabile valutare l'inserimento di strumenti necessari per garantire che non solo la parte autorizzativa, ma anche tutte le fasi successive fino alla chiusura della filiera, con la gestione dei rifiuti, siano opportunamente previste e gestite senza gravare su chi non trae giovamento dall'attività di estrazione e commercializzazione delle materie estratte. Insomma, gli interrogativi ci sono e sono critici su quella che dovrebbe essere la partecipazione effettiva della comunità territoriale, perché si tratterebbe di decisioni molto impattanti sui territori. Per questo è imperativo, o comunque dovrebbe esserlo, che ogni iniziativa legislativa tenga conto della specificità regionale, rispettando il principio di sussidiarietà e garantendo che le dichiarazioni centrali siano supportate da un dialogo effettivo e costruttivo con le Regioni. Sarebbe stato già sufficiente se nei procedimenti di rilascio dei titoli - autorizzazione al riciclaggio, trasformazione delle materie prime critiche e strategiche - fosse stato previsto un ruolo procedimentale dalla Regione interessata, così come sarebbero da chiarire le modalità di versamento dei canoni alle Regioni. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti nel tentativo di superare queste lacune. Nello specifico, per quanto riguarda il grave mancato coinvolgimento delle Regioni, abbiamo chiesto di introdurre il parere vincolante delle Regioni all'adozione delle determinazioni del Comitato interministeriale delle amministrazioni competenti sulla verifica delle istanze per il rilascio di tutti i titoli abilitativi. Abbiamo, inoltre, chiesto l'obbligo di consultare le amministrazioni regionali e locali anche per il monitoraggio strategico. tutte proposte di cui non si è colta l'importanza e che sono state, infatti, puntualmente ignorate, con buona pace del principio di leale collaborazione, che dovrebbe invece guidare l'azione del Governo. Ci sono poi anche altri elementi che ci rendono perplessi. Prima è stato citato l'ISPRA, che ha sostenuto che, con le risorse attualmente disponibili, si potrà realizzare soltanto una parte del programma, individuando - come detto - solo una ventina di aree sulle quaranta totali indicate dal decreto, ritenendo quindi improbabile, considerati Grazie che in Italia la mappatura sulle materie prime non è aggiornata, anzi è pesantemente datata. Quindi, sarebbe fondamentale e determinante aggiornare questa mappatura, tenendo conto e approfittando anche delle potenzialità che possono essere ricavate dalle azioni dell'economia circolare e da politiche di riduzione dei consumi, presupposto - lo ricordo perché ci crediamo - per gli investimenti sostenibili dalle aziende. Il problema vero e serio è che, se non si rallenta la produzione, saremo sempre più dipendenti dal ruolo di estrazione nei prossimi decenni - poi non si sa fino a quando, ma sicuramente non all'infinito considerati il quadro geopolitico ed economico, le difficoltà di approvvigionamento e i costi molto elevati. Perciò, investire nella ricerca e nello sviluppo di materiali alternativi rafforzerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento e promuoverebbe l'innovazione e la sostenibilità delle nostre tecnologie e delle politiche Riprendo quanto è emerso dall'Osservatorio italiano materie prime critiche energia, secondo il quale appaiono promettenti le prospettive di recupero da batterie, catalizzatori, aerogeneratori, pannelli fotovoltaici, mentre le elaborazioni di The European House Ambrosetti prevedono che nel 2040 il riciclo potrà soddisfare dal 20 al 32 per cento il fabbisogno nazionale di materie prime strategiche. Stiamo drammaticamente e colpevolmente perdendo un'occasione unica di modernizzazione a causa di un provvedimento privo di visione. Ecco perché abbiamo presentato una proposta emendativa che stabilirebbe l'attuazione di una strategia nazionale per l'economia circolare, attraverso la raccolta, lo smistamento, la circolarità dei materiali primi e secondi, fondamentali per i nostri imprenditori, per le nostre imprese. Perfino i consorzi RAEE, i riciclatori dei pannelli fotovoltaici e Confindustria, nel corso delle audizioni, hanno sostenuto l'importanza del recupero di tali materiali. Quindi, non è una nostra fantasia. Non meno preoccupanti sono gli effetti dell'attuazione del regolamento europeo riguardo la tutela ambientale. Per il permesso di ricerca non superiore a due anni non sarebbe neppure richiesta la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nella valutazione di incidenza, pur trattandosi di attività in grado di impattare in maniera significativa sugli ecosistemi. Ma è uno scherzo? Inoltre, il decreto-legge limita l'applicazione delle forme di tutela sanitaria e ambientale, segno ulteriore di non aver compreso da parte di questa maggioranza le potenzialità delle valutazioni ambientali e le le opportunità, anche economiche, di politiche orientate all'economia circolare e alla sostenibilità. Questo testo non considera che, secondo lo stesso Regolamento, la dichiarazione di pubblica utilità è subordinata al rispetto degli obblighi ambientali in materia di valutazione di incidenza relativi alle acque, alla salute, alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce. Presidente, mi esprimo anche a nome della mia Regione, la Sardegna, che ha espresso un parere fortemente contrario all'impostazione di questo provvedimento, che - lo ribadisco - esclude in malo modo le Regioni, imponendo addirittura, nel nostro caso specifico, una normativa che non rispetta lo Statuto sardo e le sue competenze in materia di sfruttamento di cave e miniere. Ecco perché, una volta che questo decreto-legge convertito in legge, la Regione Sardegna lo impugnerà davanti alla Corte costituzionale. Ricordo inoltre che il mio territorio presenta - è vero - una quantità importante di insediamenti minerari, forse senza pari in Italia; però è anche vero che questa forte densità risulta essere testimonianza di attività che ci hanno lasciato in eredità cave e miniere dismesse e rifiuti non gestiti. Questo è un altro aspetto importante da evidenziare: l'assenza nel provvedimento di una disciplina che riguardi la dismissione e il ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture impiegate Il testo in discussione enuncia anche i progetti di estrazioni minerarie in mare. Ebbene, riteniamo di dover ricordare che le aziende italiane potenzialmente interessate interessate alle estrazioni minerarie negli abissi sono prive di politiche a tutela del mare. Ci sono esempi di importanti società che negli ultimi anni hanno stretto accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali. Consigliamo l'opportunità di attendere la regolamentazione da parte dell'autorità internazionale competente, che deve regolamentare queste estrazioni minerarie. Infine, Presidente, voglio ricordare le conseguenze di natura sociale delle attività in miniere, dove lo sfruttamento e l'insensibilità totale alle condizioni ambientali e sanitarie non sono storie del passato. passato. Recentemente abbiamo ascoltato tristi storie in questo senso e anche quelle del contesto minerario potrebbero essere all'ordine del giorno. quindi vi siano metodi e norme irragionevoli, sotto il profilo istituzionale, ambientale, economico e sociale, che ci spingono a essere non soltanto critici verso questo atto, ma anche seriamente preoccupati per le conseguenze

Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge sulle materie prime critiche è un provvedimento cruciale per il futuro del sistema economico del nostro Paese e dell'Europa. il provvedimento in esame, il Governo ha inteso disciplinare in via d'urgenza un tema diventato di grandissima attualità a causa dell'instabilità geopolitica degli ultimi anni. E lo ha fatto adeguando l'ordinamento nazionale a disposizioni del nuovo Regolamento europeo sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche. Come è noto, la Commissione europea ha stilato un elenco di 34 materie prime che sono indispensabili per molti settori industriali, quali ad esempio il digitale, la difesa, la sanità, La domanda di materie prime critiche è necessariamente destinata ad aumentare nei prossimi decenni e, purtroppo, l'Italia e l'Europa sono quasi totalmente dipendenti dalle importazioni di tali materie da Paesi extraeuropei che spesso e volentieri sono nostri diretti *competitor* nel mercato globale. Pensiamo alla Cina comunista, che non solo fa concorrenza sleale alle imprese italiane, ma che rappresenta anche il più grande pericolo per la libertà e la democrazia del mondo occidentale. Ebbene - come tutti sappiamo- la Cina è il vero *dominus* mondiale delle materie prime e agisce praticamente in regime di monopolio su molte di tali materie.

Oppure basti pensare che l'Unione europea acquista il 97 per cento del magnesio dalla Cina e che le terre pesanti rare, da cui si ottengono i magneti utilizzati nelle auto elettriche, sono raffinate esclusivamente in Cina. Questa situazione di assoluta sudditanza e dipendenza nei confronti della Cina comunista rappresenta un problema enorme per l'Europa, che per troppo tempo ha sottovalutato detto pericolo. Le responsabilità di questa situazione sono chiaramente da attribuire alle forze politiche della sinistra, che in questi anni hanno governato male in Italia e in Europa e che in molti casi hanno preferito svendere il nostro patrimonio industriale alla Cina, come dimostra la scandalosa decisione dell'Europa di produrre solo auto elettriche a partire dal 2035. Allora, cari colleghi, ben venga questo decreto-legge del Governo che segna un importante cambio di passo rispetto al passato e punta a raggiungere una maggiore autonomia nel campo delle materie prime. Finalmente questo decreto mette in campo un piano di azioni strutturali, come la realizzazione di un programma nazionale di estrazione, l'individuazione dei progetti di interesse strategico e la semplificazione burocratica nella ricerca delle materie prime, senza dimenticare l'importantissimo intervento economico del Fondo nazionale del made in Italy e la possibilità di recuperare risorse minerarie dai rifiuti urbani ed estrattivi. Se pensiamo che nel sottosuolo italiano sono presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche individuate dall'Europa e che in Italia ci sono 3.000 siti da cui estrarre materie prime come litio, cobalto e nichel, si capisce molto bene quale sia la portata di questo decreto per il futuro del sistema produttivo italiano. Il provvedimento ha il grande merito di colmare un vuoto normativo, tagliare la burocrazia e soprattutto rilanciare la politica mineraria del nostro Paese. Grazie a questa legge avremo finalmente gli strumenti per riaprire le miniere chiuse da trent'anni, in sicurezza e nel pieno rispetto ambientale, riattivando un settore fondamentale per la nostra economia, che potrà beneficiare di un miliardo di euro del Fondo nazionale del made in Italy. In conclusione, gentili colleghi, grazie a questo provvedimento ambizioso e lungimirante abbiamo creato le giuste condizioni affinché le imprese italiane possano affrontare con successo la doppia sfida della transizione ecologica e digitale, ben consapevoli che l'accesso alle materie prime rappresenta un elemento essenziale per la nostra conversione si inserisce pienamente nel solco di altri provvedimenti adottati dalla maggioranza e dal Governo di centrodestra che dimostrano in maniera chiarissima la nostra volontà di tutelare e promuovere lo sviluppo delle imprese e del mondo produttivo italiano. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare con forza e determinazione per garantire lavoro, sviluppo e benessere al nostro Paese, ai nostri cittadini e alle nostre imprese.

onorevoli senatori, cominciamo fornendo alcuni numeri che ci fanno capire di cosa stiamo parlando. L'Unione europea acquista il 97 per cento del magnesio in Cina; le terre rare pesanti, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, sono raffinate esclusivamente in Cina; il 63 per cento del cobalto mondiale utilizzato nelle batterie è estratto dalla Repubblica Democratica del Congo; il 60 per cento è raffinato in Cina.

Noi veniamo da un periodo in cui a un certo punto, nella nostra vita come cittadini europei e come cittadini del nostro Paese, abbiamo impattato, per la prima volta, con cosa significa non avere a disposizione materie prime e materie prime critiche, come quelle di cui stiamo parlando. Durante la pandemia, il crollo e il blocco delle materie prime ci hanno visto in difficoltà, ad esempio per quanto riguarda tutto il settore della chimica, per la produzione dei farmaci, ma anche per l'approvvigionamento dell'*automotive* o delle materie che ci servono per adeguare le nostre tecnologie al sistema mondiale (quindi tutta la trasformazione digitale e *green*).

alla prospettiva - dobbiamo ovviamente scongiurarla e per questo stiamo parlando di questa materia - che ci possano essere nuove situazioni di criticità, legate a fattori geopolitici o a pandemie, che possano farci trovare in una difficoltà di approvvigionamento delle materie che tengono insieme il nostro sistema di difesa, il nostro sistema tecnologico, il nostro sistema industriale, i nostri sistemi sanitari e le tecnologie intorno alle quali abbiamo costruito le nostre vite. A torto o a ragione, questa è la realtà in cui ci troviamo.

ad esempio in Cina, e poi le abbiamo pagate il doppio. L'altro grande tema è il riciclo di quella grande miniera a cielo aperto che sono i nostri scarti industriali e i nostri rifiuti tecnologici, che spesso entrano in mercati paralleli (mercati neri), che vengono rubati

avendo il tempo di intervenire in un dibattito parlamentare nelle Commissioni di competenza, che non è soltanto quella delle attività produttive, ma ci sono l'ambiente, la salute, i termini legati alle Regioni e al coinvolgimento dell'istruzione e della ricerca. Invece

perché spetta a loro la funzione di tutela del Parlamento e di ciò che rappresenta rispetto alle comunità che qui sono coinvolte. *(Applausi)*. Il secondo elemento - lo dico con un certo stupore è che dall'impianto tecnico del decreto, sia sul punto unico di contatto, sia sul nuovo Comitato che viene istituito presso il Ministero, sia sulle procedure di autorizzazione della valutazione viene esclusa la partecipazione delle Regioni. Badiamo bene: qui non siamo in materia di autonomia differenziata, ma questa è una materia già delegata alle Regioni.

tolgono funzioni e competenze già in capo alle Regioni. È una contraddizione - voglio dirvi - non soltanto dannosa, ma anche inutile. Nell'esperienza che tutti noi abbiamo avuto con le grandi infrastrutture pensiamo alle autostrade, ai treni, alle dighe o alla TAV - se non hai gli enti locali al tavolo, tu Governo puoi fare tutti i decreti che vuoi, ma il provvedimento non lo porti a casa In un Paese che non fa più estrazioni minerarie da trent'anni, il Piano qui predisposto richiede una complessità di interventi sui territori invasiva. Voi pensate che si possa andare avanti con questi obiettivi, per quanto strategici, senza aver avuto un coinvolgimento al tavolo decisionale, in questo famoso punto unico di contatto, degli enti territoriali, dei sindaci, dei Presidenti di Regione? Pensiamo alla Sardegna, che è il più grande bacino minerario in Italia, tra l'altro quello che ha anche un'esperienza ancora attiva. Che cosa significa prendere decisioni di questo tipo senza poter sapere com'è composto un territorio, qual è l'impatto ambientale? Su quello che ambientale? Su quello che è un decreto-legge che dovrebbe affrontare una questione strategica di interesse nazionale, questo è - permettetemi - un errore strategico di prospettiva, di capacità di prevedere i problemi e poterli risolvere. Si parte già con il piede del conflitto: è un errore da penna Un altro aspetto importante che viene trascurato in questo decreto-legge è legato alla parte delle manovalanze. Noi non abbiamo maestranze minerarie, non si fanno più scavi in Italia. Quanti anni sono? Sono decenni. C'è un'unica università in Italia che se ne occupa, che è il Politecnico di Torino e ha una scuola mineraria, dove ci sono pochissimi iscritti, quasi tutti stranieri. È evidente che in un impianto come questo c'era e c'è la necessità anche di costruire le competenze e le risorse umane per fare una nuova filiera strategica di cui noi abbiamo bisogno. Mi avvio a concludere con l'ultimo punto, Presidente, che è quello del riciclo, è appena accennato in questo provvedimento, come ho detto nelle premesse. Noi sul riciclo, con un investimento di 500 milioni - come ci hanno detto durante le audizioni - potremmo andare oltre gli obiettivi previsti entro il 2040, cioè potremmo raggiungere cento del nostro fabbisogno ed estrarre una quantità di materie prime critiche enorme e nello stesso tempo avviare una catena virtuosa che ci permette anche di gestire il ciclo dei rifiuti come una risorsa e non soltanto come un costo ambientale, o un peso nelle nostre strutture e nelle nostre vite.

parere contrario su tutti gli emendamenti.

riguarda l'articolo 1, nel raggiungimento degli obiettivi - come diceva giustamente la collega Lorenzin - un tema estremamente importante è quello del riciclaggio delle materie prime. Riteniamo che i nostri emendamenti al propedeutici a garantire e migliorare il sistema di recupero delle materie prime. È inoltre necessario che, accanto a questa norma, sia applicata anche tutta una serie di modifiche alle normative esistenti, visto che di fatto rendono impossibile per un singolo cittadino o una piccola impresa poter intervenire

fondamentale nel garantire la raccolta differenziata del rifiuto urbano, deve essere data la possibilità di estendere tale attività anche alla gestione dei piccoli rifiuti delle imprese, di migliorare ed elevare la raccolta differenziata. Ci deve però essere un pari incentivo, altrimenti aumentano i costi e si disincentivano le persone, le famiglie e le imprese alla raccolta,

per velocizzare l'autorizzazione - non c'è una VIA, neanche a pagarla oro - ci stupisce il parere contrario a un emendamento che non dice altro che riaprire siti dismessi, che avevano già ottenuto tutte le autorizzazioni e che erano stati dismessi perché non più considerati economici. Invece di ripristinare dei siti dismessi, si vanno a cercare terre rare in tutto il resto del Paese, magari in zone che non sono proprio felici di veder aprire delle miniere a cielo aperto, perché magari, nel frattempo, sono diventate zone turistiche, zone di attrazione, zone di tutela. Quindi, ci sembra veramente buffo che, invece che tornare in una zona dove tutto questo potrebbe avvenire con maggiore facilità, si decida di non tornare su luoghi che avevano già avuto un'attività estrattiva in origine. Per questo abbiamo presentato questo emendamento. Vedo che il collega Martella ne ha presentato

chi deve estrarre deve anche impegnarsi a ripristinare le condizioni dal punto di vista ambientale, predisponendo un piano che vada in questa direzione. Non si capisce chi lo dovrebbe fare.

parere contrario su tutti gli emendamenti.

«ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per avviare attività di riqualificazione e formazione dei lavoratori del comparto minerario».

a condizione che siano accolte le seguenti modifiche: sopprimere tutte le premesse sino al dispositivo ed eliminare dall'impegno le parole: «nel primo provvedimento utile» e le parole: «sui principali mezzi di comunicazione».

È chiaro ed evidente che oggi molte Regioni, Comuni e Province si trovano a fare i conti con i recuperi ambientali, anche dal punto di vista paesaggistico, di siti dismessi.

caratterizzazione dei siti ai fini della bonifica e anche a dover emettere le ordinanze. E chi sa di amministrazione sa benissimo che cosa avviene quando si fanno le ordinanze: se il soggetto adempie, deve adempiere l'ente locale. Molto spesso si parla di interventi straordinariamente elevati, che pertanto non sono sostenibili dagli enti.

Signora Presidente, l'inconcludenza di questo decreto-legge la si evince dal parere contrario a un ordine del giorno; neanche a un emendamento, che riapre la possibilità di votare il provvedimento alla Camera, ma a un ordine del giorno, che, da tre legislature a questa parte, mi hanno insegnato più o meno non si nega a nessuno. Si tratta di un ordine del giorno che prevede banalmente di ampliare le materie prime

dalle telecomunicazioni alla transizione ecologica. Non si capisce perché, visto che questo provvedimento serve ad attuare una filiera italiana, non lo si fa su tutti i metalli pesanti che servono per questa filiera. Estraiamo "a muzzo": qualcuno sì e qualcun altro no. Come tale, questo è un decreto non serio, perché, se si vuole creare una filiera, si prendono in mano tutti i metalli che noi abbiamo e che servono

questo è un decreto *maquillage*, che non serve né alla transizione ecologica, né alla filiera italiana. Serve per far vedere all'Europa che ce ne siamo fregati della loro direttiva e che abbiamo fatto di testa nostra; lo si vede dai materiali che andiamo a estrarre, così, random.

Signora Presidente, siamo quasi giunti al termine della votazione di questo provvedimento. Tanti emendamenti puntavano proprio l'attenzione sul riciclo e, quindi, sulla necessità per essere autonomi da queste materie

Deve restare agli atti quanto fondamentale sia puntare sul riuso e anche sui fondi che devono essere stanziati a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati anche alla tracciabilità e quindi alla possibilità di allungare al massimo la vita di tutto ciò che è progettato e che utilizza queste materie critiche. promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori, in modo da dare una vita a queste materie critiche che sia

perché parliamo di risorse fondamentali per la nostra economia, che influenzano settori chiave come l'energia, l'*automotive*, la tecnologia, il campo mediatico, la difesa e l'aerospazio. È proprio dalla loro rilevanza per il sistema produttivo e, al contempo, dai possibili rischi delle forniture che queste materie prime le possiamo definire critiche. Sono materie prime infatti esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, a causa molto spesso dell'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi. non solo una forte dipendenza dall'estero, ma anche e soprattutto esposizione alle forti tensioni internazionali. Quello delle materie prime critiche è infatti un tema che inevitabilmente ci porta a riconsiderare la dipendenza della nostra Nazione dalle importazioni di queste materie da Paesi extra-UE, che molto spesso sono politicamente ed economicamente instabili, tanto che abbiamo anche assistito ad interruzioni e rallentamenti nella catena degli approvvigionamenti, specie in diretta conseguenza dei recenti eventi geopolitici. Questa dipendenza - è inutile dirlo - impatta negativamente su importanti settori strategici come il settore dell'energia, se pensiamo che la produzione di energia rinnovabile da pannelli solari, turbine eoliche e batterie e batterie richiede materiali critici come il litio e il cobalto. Non avere una produzione interna aumenta i costi e rende l'Italia vulnerabile alle fluttuazioni del mercato, ma soprattutto ci rende fortemente dipendenti dalla Cina *in primis*, che riesce a produrre prodotti finiti a basso costo. impatta sul settore della mobilità, perché la transizione verso i veicoli elettrici dipende fortemente dalle batterie agli ioni di litio. Materie prime scarse, dunque, equivalgono a limitare la produzione di veicoli elettrici, ad aumentare i costi per i produttori italiani, a favorire la delocalizzazione e, infine, a compromettere la nostra competitività nel mercato globale. Ancora, questa scarsità di materie prime strategiche può impattare negativamente sull'industria tecnologica ed elettronica (se pensiamo alla componentistica dei nostri *smartphone* e PC), sul settore della difesa e dell'aerospazio, come pure sul settore manifatturiero. Per questo motivo era urgente ridurre la dipendenza e rafforzare l'autonomia del nostro sistema economico e produttivo. produttivo. Il decreto-legge in esame, dunque, va proprio nella direzione di risolvere il tallone d'Achille della dipendenza europea dalle materie prime fondamentali per l'industria, rappresentando al tempo stesso un tassello molto importante nel quadro di iniziative che il Governo Meloni ha messo in atto per garantire al nostro Paese di affrontare a testa alta le principali sfide economiche, climatiche ed energetiche. Un provvedimento che innanzitutto ci consente di recuperare una parte importante dell'industria italiana, quella mineraria, ferma da decenni, in un periodo di tempo in cui il mondo e altri Paesi europei non sono stati a guardare mentre in Italia si è passati da circa 3.000 siti minerari, censiti negli anni precedenti, agli attuali

energetica e, come dicevo, ben 3.000 siti da cui poter estrarre materie prime critiche (in particolare litio, cobalto, barite, berillio, nickel, tungsteno, rame, zinco), si capisce perché e soprattutto quanto sia importante questo decreto-legge. Non è certo un segreto che sull'Appennino ligure-emiliano, sulle Alpi occidentali, nel mio Trentino, in Carnia e in Sardegna si può trovare il rame, oppure che giacimenti di tungsteno esistano in Calabria, in Sardegna e sulle Alpi. In Piemonte e in Sardegna si trova il cobalto, in Toscana la magnesite, mentre il litio è stato scoperto nei fluidi geotermici di Toscana, Lazio e Campania. Abbiamo un patrimonio inestimabile di materie prime critiche che, proprio come una bella addormentata nel bosco, deve essere risvegliato. Questo decreto-legge, come dicevo, mira proprio in questa direzione e pone le basi per riattivare quei processi di ricerca, coltivazione, estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, perché quello che vogliamo fare è essenzialmente dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese; rafforzare la *governance*

di sostenibilità. Per fare questo, colleghi, dobbiamo ragionare in termini di discontinuità rispetto al passato, se vogliamo intraprendere la strada dell'innovazione e della sostenibilità. Non un passo indietro, quanto piuttosto molti passi avanti sulla via del rafforzamento e dello sviluppo economico sostenibile per l'ambiente e per la società. Sotto questo aspetto, lasciatemi dire, fa sorridere l'ipocrisia dei soliti fautori del no a tutto o di coloro che, con una mano, si oppongono a qualsiasi attività estrattiva nel nostro Paese, anche delle materie prime critiche necessarie alla decarbonizzazione, e, con l'altra mano, invocano l'applicazione di una linea politica che sottostà completamente a questo tipo di dipendenza, glissando totalmente sulle condizioni disumane con cui vengono estratte nei Paesi in via di sviluppo, in Africa soprattutto e ad opera spesso di bambini. Colleghi, è ora di svegliarsi e di guardare in faccia la realtà. Abbiamo la Cina, da un lato, che stringe accordi di produzione mineraria con settanta Stati e, dall'altro, abbiamo l'Unione europea che è quasi ferma al palo, in clamoroso ritardo. In questo scenario, l'Italia, la nostra Nazione, anziché aspettare Godot, intende rispondere a chiare lettere con questo provvedimento. Un provvedimento capace di dare pronta risposta ai problemi di approvvigionamento e dotare la nostra economia di un sistema più efficiente e resiliente, basato sui principi del libero mercato e della concorrenza, per raggiungere anche questa sovranità tecnologica delle reti e delle infrastrutture. Vedete, colleghi, è proprio da questo fondamentale snodo che passano, non solo la resilienza e la crescita

danni che sta creando la sinistra europea con l'accelerazione *green*, tutta infarcita di ideologia ma che, di fatto, ha dimostrato di non essere sostenibile dal punto di vista sociale ed economico per il nostro Paese, per le imprese e per le nostre famiglie. Politiche industriali, quindi, il che significa nuove *partnership* strategiche con altri Paesi. Da questo punto di vista, il successo del recente incontro del presidente Meloni con il presidente Xi Jinping è è la plastica dimostrazione di come una cooperazione equilibrata, mutualmente vantaggiosa, basata sulla reciproca fiducia, possa rafforzare la nostra posizione economica, la nostra credibilità, garantendo la competitività e l'innovazione del nostro sistema industriale. Signor Presidente, solo con un approccio pragmatico e concreto potremo ridurre la nostra vulnerabilità e costruire un futuro più resiliente e sostenibile. È l'approccio che questo Governo, grazie al sostegno sempre più convinto e autentico degli italiani, dimostra di avere con i fatti, non con le chiacchiere. Rendiamoci più indipendenti, più forti, più resilienti. Puntiamo allo sviluppo e alla crescita della nostra Nazione. L'approvazione di questo provvedimento è un passo importante in questa direzione.

emendamenti di fatto non letti, perché bocciati nel giro di mezz'ora, con votazioni velocissime, senza neanche possibilità di esaminarli, ordini del giorno anche quelli letti più o meno frettolosamente. Ieri la collega Tubetti ci ha dato una lezione di politica: l'opposizione pensa alle vacanze, a stare a Capalbio e ad una vita agiata, noi facciamo il bene del Paese. Voi, che siete persone scollegate dalla realtà, non capite che la rete ferroviaria italiana non verrà bloccata perché il ministro Salvini non sa fare una programmazione e rispettare l'unica settimana di vacanze che gli italiani normali, non quelli di Capalbio, fanno, cioè quella di Ferragosto. No: è RFI È il gestore che ha deciso il blocco della linea. Io ho abbastanza sorriso al fatto che la concretezza della politica si appresti a dire che questo

nell'attività di impresa privata. Per quanto riguarda invece le proprie partecipate, lì non tocchiamo boccino *(Applausi)*; nonostante la nomina del presidente e dell'amministratore delegato avvenga per via governativa e parlamentare, lì possono fare tutto quello che vogliono, noi ci occupiamo delle Olimpiadi francesi. Evidentemente eravate talmente distratti dalle Olimpiadi che avete fatto un decreto assolutamente inutile. Lo dico con molta simpatia alla collega Biancofiore, alla quale mi lega veramente una simpatia personale;

come ha dimostrato il mio ordine del giorno, non si va neanche alla ricerca di tutte quelle terre rare che servono per la transizione ecologica e per tutto quello che l'Italia sa fare, ma viene deciso così prioritariamente di cercarne alcune e di lasciarne indietro altre.

Regioni. Avete votato l'autonomia differenziata dicendo che serviva per il Paese. Noi di Italia Viva, come opposizione, non siamo d'accordo su questo, tanto è vero che stiamo raccogliendo le firme per il *referendum*. Fate poi un provvedimento sulle terre rare

sono i soggetti interessati a dare l'autorizzazione. Delle due l'una: o l'autonomia differenziata, in questo caso addirittura il Titolo V così come è, senza un ulteriore passo avanti, da rispettare o se ogni volta che invece bisogna semplificare, si va verso una centralizzazione, allora la pensate come noi. Mi spiace non avere i moduli per farvi firmare il *referendum* contro l'autonomia differenziata perché questo decreto lo è.

alla narrativa continua fatta da questa maggioranza e dalla Presidente del Consiglio. Si dice che finalmente noi siamo determinanti in Europa, prevediamo un decreto che non è collegato con un regolamento europeo. Si dice poi che finalmente siamo determinati nel mondo. Spero che quando siete andati in Cina, abbiate fatto un accordo con la Cina sulle terre rare. Concludo

Il gas è importantissimo, ma tutto quello che è il futuro lo lasciamo giustamente, per i rapporti politici che avete, ai russi e ai cinesi. Mi sembra la degna conclusione della vostra priorità per il Paese. quindi, che ci fosse una frase del tipo: con il Piano Mattei prevedremo degli accordi bilaterali con i Paesi per estrarre quelle materie prime rare che servono

primo in Europa e vorrebbe, per quanto riguarda le materie rare, essere ancora più avvantaggiato. Sicuramente ci sono degli impianti da creare e il PNRR, approvato con il ministro

fare un primo scavo in uno dei territori elencati nella dichiarazione di voto della collega Biancofiore, non solo troverete i comitati del no, ma troverete un ricorso alla Corte costituzionale delle Regioni che purtroppo verrà vinto. Per questi motivi, perché è così inutile da essere imbarazzante, voteremo convintamente contro il

innanzitutto per un aspetto che abbiamo più volte sottolineato, cioè il ruolo delle Regioni e degli enti locali. Pertanto, nonostante l'articolo 1 preveda che le disposizioni del decreto-legge vengano attuate nel rispetto degli attuali statuti e delle norme in attuazione, le Regioni

viene loro richiesto un parere che non è affatto vincolante. Avete infatti riportato al livello di Governo centrale alcune delle competenze regionali proprio in materia di programmazione territoriale, disattendendo al principio di collaborazione tra Regioni e Governo. Si rischia quindi di determinare un vero e proprio scontro istituzionale su questo terreno. Devo dire che non capisco più dove volete andare. Da una parte, ci dite che volete l'autonomia delle Regioni e dall'altra centralizzate i poteri nello Stato. in questo provvedimento come in altri. Ma se vi siete pentiti di aver approvato l'autonomia differenziata, allora venite con noi a raccogliere le firme per il *referendum*, c'è posto anche per voi, anche se abbiamo già raggiunto il *quorum* richiesto. Anche rispetto alle modalità con cui autorizzate i procedimenti, ci sono state critiche persino dai responsabili della direzione dei Ministeri sia del made in Italy, sia dell'ambiente, perché non è chiaro l'*iter* da seguire, quindi c'è il rischio di altri cortocircuiti che possono creare difficoltà, anche se voi in questo momento siete fermi sul fatto di voler portare avanti queste disposizioni, tra l'altro attraverso un decreto-legge, quando invece abbiamo sottolineato più volte come sarebbe stato più adeguato seguire procedimenti legislativi differenti, che coinvolgessero maggiormente non solo il Parlamento, ma anche gli enti territoriali, magari attraverso la Conferenza Stato-Regioni. poi il fatto che, per raggiungere i tempi previsti di questo decreto, che sono estremamente stretti per alcune cose, come ha sottolineato anche l'ISPRA, dato che entro marzo del prossimo anno si dovrà definire una carta, bisognava prevedere, ad esempio, l'assunzione delle persone, perché ci sono delle forti criticità. L'ISPRA in audizione ha sottolineato un dato molto preciso,

ormai abituato a cambiare modalità, smonta e rimonta strutture esistenti sostituendole con altre, ovvero sostituendo i componenti, cioè cercando ogni occasione utile per rimediare qualche poltrona in più, questa è l'unica spiegazione, perché non si capisce per quale ragione quel tavolo A leggere bene questo decreto, sembra che il tema delle materie prime critiche sia stato solo un pretesto per creare organi di dubbia efficacia per mantenere i poteri all'interno della stessa maggioranza. Un decreto-legge non può essere lo strumento idoneo ad affrontare un tema così complesso

nella logica sempre di far da sé contro una parte e contro l'altra, rischiamo di rimanere da soli con poche cose attaccate. In conclusione, avete presentato un decreto-legge sgangherato che qua e là forse è utile per assicurare qualche posto a qualche vostro amico, ma il provvedimento alla fine, nel metodo e nel merito, non ha sostanza e non può trovarci d'accordo e quindi voteremo contro.

membri del Governo e colleghi, le fondamenta del nostro modello economico sono rappresentate dalla capacità di trasformare le risorse naturali prese dal nostro ecosistema in prodotti e il nostro modello economico esiste grazie alle materie prime. Il capitale naturale, però, è un capitale critico, perché è finito. Abbiamo una serie di *stock* di minerali che non possono essere rinnovati quando si esauriscono. Non resta dunque nulla per le generazioni future. I giacimenti non sono eterni e le quantità disponibili si esauriscono, dunque conviene iniziare a trovare alternative all'uso di alcune materie e creare condizioni ottimali per il riciclo e il riuso. Le materie critiche sono ancora più importanti; sono contenute nei nostri cellulari e nelle tecnologie innovative, come i pannelli fotovoltaici, e nel sistema di trasporto elettrico. Sono essenziali per le batterie, utilizzate come sistemi di accumulo per potenziare l'energia rinnovabile. Le abbiamo sempre usate nel tempo, solo che ora ci siamo resi conto che sono limitate e, con una popolazione in aumento a livello mondiale, con ogni individuo che possiede un cellulare e almeno un televisore, bisogna correre ai ripari. In Europa, come in Italia, non ci sono queste risorse nel sottosuolo, non ci sono quei minerali. Per questo il Governo decreta con urgenza: altro giorno, altro decreto-legge. Ma oggi, più che mai, siamo al cospetto di un decreto-legge che contiene tanti paradossi e l'irragionevolezza normativa di questo provvedimento investe tanto gli aspetti di merito quanto quelli di metodo. Partiamo dal fatto che non si fa distinzione tra le materie prime, quindi tutte vengono trattate allo stesso modo, a prescindere dalla difficoltà di estrazione o dal rischio di depauperamento. Una volta accertato che l'approvvigionamento delle materie prime critiche è fondamentale per la nostra economia, è corretto chiedersi, e mi chiedo, Presidente: se non abbiamo miniere, ma una capacità elevata di effettuare il riuso e il riciclo e quindi applicare i principi fondamentali del modello di economia circolare, perché in questo provvedimento, in cui avremmo dovuto dotarci di opportuni strumenti tecnici e normativi, volti a perseguire un modello di economia realmente *green* e circolare,

Non si comprende, poi, la linea seguita dal Governo, che da un lato continua a promuovere leggi accentratrici, come in questo caso, mentre, dall'altro, consente alle Regioni di chiedere maggiore autonomia in tante materie di interesse strategico nazionale, pensate un po', anche nella salvaguardia delle materie prime critiche. Quindi avete pensato bene di salvaguardare un interesse unitario nazionale avallando una frammentazione normativa, sapendo che è cosa impossibile. E, in piena consapevolezza, lo avete messo nero su bianco in questo decreto-legge. mentre, grazie alla scellerata legge sull'autonomia differenziata, le Regioni potranno chiedere l'autonomia e la competenza in 23 nuove materie, questo decreto-legge crea un punto unico nazionale di contatto e accentra le competenze in capo al Ministero dell'ambiente, il grande assente. Sì, Presidente, ci si chiede infatti come sia stato possibile assegnare nuove funzioni al dicastero, senza il coinvolgimento del procedimento legislativo. Forse è la dimostrazione del peso del ministro Urso nella maggioranza, tale da superare anche la ripartizione delle competenze ministeriali. Il Ministero dell'ambiente, però, ha già annunciato l'adozione di un proprio provvedimento. Insomma, decretazione di urgenza e lotte intestine incombono sulla sorte industriale del nostro Paese. Dall'articolato sembra, infatti, che il tema delle materie prime critiche sia stato solo un pretesto per creare organi di dubbia efficacia e per un riparto di potere all'interno della maggioranza. Sul tema delle materie prime critiche è stato da poco emanato un regolamento europeo, il Critical raw materials act, un atto già esecutivo in tutti gli Stati membri, nato per fornire una strategia chiara per affrontare l'accesso alle materie prime critiche. Esso si pone come traguardo il raggiungimento dell'obiettivo nel 2030. Contiene, però, numerose deleghe alla Commissione europea e sarà, quindi, integrato nel tempo. Esso ha attribuito molta importanza al recupero e al riciclo di materie prime seconde, all'*end of waste*, e solo per ultimo ha menzionato l'estrazione di materie prime. A questo punto mi domando e vi chiedo: qual è la *ratio* di questo provvedimento, Presidente? Perché la decretazione d'urgenza per l'ennesimo decreto-legge Perché non rispettare la scaletta intelligente fornita dall'Europa? andrebbe anche incontro alle richieste delle imprese, che, nonostante un Governo ostile ai temi della transizione ecologica e dell'economia circolare, continuano a rendere l'Italia uno dei Paesi più avanzati e innovativi in questo settore. Soltanto chi, come questa maggioranza, ha una visione limitata può pensare che si tratti di temi estranei al decreto in esame. Basterebbe poco per comprendere che la tutela delle materie prime critiche parte proprio dal contenimento del loro utilizzo e dal loro riciclo. Vogliamo che le nostre imprese siano competitive sui mercati internazionali? Bene, allora lavoriamo per sostenere l'*ecodesign* sistemico e implementiamo misure per creare professioni nuove, necessarie alle imprese che non trovano personale qualificato nei settori *green* e digitale. I licei del made in Italy sono stati un fallimento perché non attrattivi con insegnamenti non innovativi. Il MoVimento 5 Stelle, a tal proposito, ne aveva emendato il testo, suggerendo l'inserimento di insegnamenti come la merceologia, i cicli di produzione, la valutazione del ciclo di vita (il famoso *life cycle assessment*) la contabilità ambientale. Questo è necessario insegnare ai tecnici del made in Italy per consentire loro di calcolare la sostenibilità e migliorare i processi, i prodotti e i servizi forniti alle nostre imprese,

un'economia che verrebbe fortemente danneggiata dall'apertura di miniere estrattive sia su terraferma, che in mare. Per cosa, poi? Per raschiare il fondo del barile, perché in realtà non abbiamo un granché. È lo stesso errore fatto dal Governo con le autorizzazioni alle trivelle in mare: poca materia, che coprirebbe il fabbisogno interno solo per un anno. Le concessioni sono però in mano ai privati (e non al pubblico), che possono decidere di vendere la risorsa estratta al miglior offerente. Con i minerali estratti in Italia avverrà la stessa cosa: i privati venderanno al miglior offerente in Italia. Sapete cosa resterà? Il danno ambientale, che pagheremo poi noi con le nostre tasche, la nostra salute danneggiata e un territorio deturpato che non sarà più attrattivo.

Incentivare l'economia circolare, quindi, significa non solo abbattere le emissioni di gas climalteranti, ma anche diminuire l'uso di capitale naturale e - ancora - creare posti di lavoro, una nuova occupazione che scaturisce dalla creazione della filiera inversa, chiamata così perché, inversamente all'economia lineare che si chiude con un rifiuto da eliminare in discarica o incenerire, continua con una serie di processi (raccolta, riuso, riciclo meccanico e chimico), creando creando materie prime e seconde che rientrano in azienda come *input*. Questo Governo non segue purtroppo la visione circolare. Riaprire e dare concessioni per estrarre materie prime e non porre attenzione all'*urban mining* significa andare nel senso opposto. Si continua con il modello di economia lineare.

di processo e prodotto ed effettueranno il sorpasso delle imprese italiane, non supportate da adeguati incentivi e normative, nonostante le loro grandi capacità imprenditoriali. Un'ulteriore gravissima criticità consiste poi nel non aver effettuato un bilancio della risorsa acqua. Abbiamo devastanti problemi di siccità che non riusciamo a combattere. Sapete quanta acqua serve per estrarre minerali? Decine di milioni di litri al giorno. E da dove la prenderemo? Ma, soprattutto, a chi andremo a toglierla? Infine, non una parola sul *database* pubblico che dovrebbe consentire la geolocalizzazione e la visualizzazione di risorse o materiale riciclabile nelle nostre città (il famoso *urban mining*). Pare che si affronterà tutto questo in un secondo provvedimento, ma l'approccio sistemico insegna a valutare le interazioni fra i sistemi per poter correggere le derive e cavalcare la complessità. In conclusione, alla luce di quanto esposto, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

oggi un provvedimento che interessa tutte le fasi della filiera delle materie prime critiche (dalla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione, fino al riciclo) e si concentra in particolare sulla semplificazione delle procedure autorizzative. Infatti, i permessi verranno rilasciati in un tempo massimo di diciotto mesi per le attività estrattive e di dieci mesi per quelle volte alla lavorazione e al riciclaggio. A occuparsi del monitoraggio delle catene di approvvigionamento di queste materie prime critiche, delle loro scorte e delle esigenze di fornitura delle aziende sarà un apposito comitato tecnico, chiamato appunto Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche, che verrà fatto confluire all'interno del Mimit. Ogni tre anni il comitato dovrà presentare un piano nazionale integrato delle materie prime critiche e quindi un documento contenente gli obiettivi, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili. All'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sarà invece affidata l'elaborazione di un programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con la relativa mappatura dei minerali strategici presenti sul territorio italiano. Parliamo di un potenziale minerario dell'Italia attualmente ignoto, perché le esplorazioni degli elementi critici sono state interrotte decenni fa, con la chiusura di quasi tutte le miniere. Ma adesso possiamo finalmente guardare nuovamente al futuro, perché il Fondo nazionale del made in Italy, partecipato dal MEF, verrà modificato proprio per includere nel suo campo di applicazione anche le attività legate all'estrazione e alla trasformazione delle materie prime critiche. Le risorse del fondo (lo stanziamento iniziale è pari a un miliardo di euro) potranno venire incrementate anche con risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni; è prevista anche la possibilità di investire in strumenti di rischio emessi da società di capitale con sede in Italia, non operanti chiaramente nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Già un anno fa questo Governo, ricordando gli obiettivi europei sull'estrazione delle materie prime critiche per ridurre la dipendenza eccessiva dall'estero, in particolare dalla Cina (come hanno ricordato molti colleghi prima), aveva sottolineato la necessità per l'Italia di aprire nuove miniere. Trent'anni fa l'Italia era un grande Paese minerario. Abbiamo chiuso tante miniere per svariate ragioni; ora dobbiamo riaprirle e magari ne apriremo altre ancora, perché non ci spaventa il futuro e soprattutto non ci ferma l'ideologia. I giacimenti italiani di litio, un metallo essenziale per le batterie di tutto ciò che usiamo quotidianamente, già si concentrano attualmente - come ricordava il mio collega Bergesio prima in discussione generale tra Toscana, Lazio e Campania, in particolare nell'area a Nord di Roma. Quelli di cobalto, un altro metallo utilizzato negli accumulatori, benché si stia cercando di sostituirlo, sono in Piemonte, a Punta Corna, ma anche nel Lazio settentrionale. Il Sud della Sardegna contiene terre rare per i magneti dei veicoli elettrici e la fluorite per l'alluminio; il rame per i cavi elettrici si trova in Veneto, in Lombardia e in Toscana, il manganese per le batterie e per l'acciaio in Abruzzo, Calabria e Sicilia. Il buon Dio quindi - è l'ennesima prova - ha regalato all'Italia tutto. Troppo spesso, però, è mancato il coraggio di trasformare in risorsa ciò che di prezioso abbiamo. Il segmento della trasformazione delle materie prime in prodotti intermedi e finiti, come i magneti in terre rare, è infatti quello a maggior valore aggiunto, nonché il più cruciale, in quanto direttamente connesso alle altre applicazioni industriali. In altre parole, come di solito non si utilizza direttamente il petrolio greggio, ma i derivati della raffinazione, come la benzina, così non si utilizzano i minerali grezzi, bensì quelli lavorati. Questo provvedimento rappresenta una piccolissima rivoluzione, l'inizio di un percorso, perché va a sfidare i nuovi pagani, che credono e fanno credere che basterebbe non usare più il petrolio e il gas per porre fine alle estrazioni del sottosuolo. Evidentemente pensano, questi signori, che l'energia solare e/o eolica sia creata senza creata senza scavare né sporcare. In altre parole, la vera minaccia alla crescita di questo Paese è l'eccesso dell'ambientalismo, che, tra le tante cose, ha modificato nell'opinione pubblica anche il concetto di risorsa come definita dalla natura. Se così fosse, la quantità di risorse dovrebbe essere un dato conosciuto e misurabile; ma non è così, anzi la storia insegna che le risorse sono andate sempre diversificandosi e moltiplicandosi. Se pensiamo ai miracoli, possiamo vedere che nel ventesimo secolo le riserve conosciute di tutti i minerali si sono sono moltiplicate e i costi sono diminuiti in misura ben maggiore rispetto all'aumento della popolazione, che pure nel giro di un secolo si è quadruplicata.

cento. La verità è che l'elemento essenziale che fa di qualsiasi cosa una risorsa è il lavoro dell'uomo. Dietro qualsivoglia minerale c'è un lavoro di esplorazione, estrazione e lavorazione che ne dà valore e questo vale anche per le risorse più naturali e comuni. Un esempio? L'acqua. Nessuno si lava o beve dalle sorgenti; l'acqua arriva in casa grazie al lavoro di chi ha ideato e realizzato acquedotti, gli impianti di potabilizzazione, Si parla solo di risorse consumate, ma mai una parola su come vengono prodotte. A definire la risorsa non è la natura, ma è l'uomo e la sua capacità, è la sua creatività di usare gli elementi della La vera risorsa è dunque proprio l'uomo e come Lega abbiamo sempre guardato a questo per strutturare misure che avessero cura del Creato, producessero prospettive non ideologiche per il futuro e rappresentassero una risposta concreta e reale per un mondo che, naturalmente, cambia.

colleghe senatrici, colleghi senatori, signora rappresentante del Governo, ci troviamo oggi nuovamente a votare un testo chiuso, un decreto-legge che non solo limita il ruolo del Parlamento, ma mortifica anche la qualità della nostra legislazione. Rispetto a un tema così delicato e complesso ci saremmo aspettati ben altra attenzione, ben altra disponibilità. Sarebbe stato necessario un confronto reale e proficuo, che permettesse un doveroso approfondimento. Infatti noi, come Gruppo parlamentare, già a febbraio di quest'anno avevamo presentato una mozione sul tema delle materie critiche e strategiche: un tema cruciale per la competitività del nostro Paese, sia in termini economici, sia per le complesse evoluzioni geopolitiche di questo momento storico, sia per affrontare in maniera adeguata le transizioni ecologiche e digitali. Il fatto è che ormai questo Governo in due anni ha mostrato moltissimi limiti, ma è proprio sulle politiche industriali che ha fallito maggiormente. Non lo diciamo solo noi,

Invece noi pensiamo che l'Italia sia e debba rimanere un Paese industrializzato e un Paese *leader* a livello europeo, ma con voi è sempre più evidente il rischio di perdere ulteriormente competitività sui mercati internazionali. Com'è noto, il decreto-legge in esame cerca di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, che ora è di competenza regionale. Lo fa richiamandosi ad un regolamento europeo recentemente approvato, nell'aprile di quest'anno, che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie critiche. Questo regolamento - voglio ricordarlo ai colleghi della maggioranza - è uno dei pilastri del *green deal* europeo, un modello di sviluppo che due dei principali partiti di questa maggioranza hanno recentemente contrastato - è bene ricordarlo - votando contro la presidenza von der Leyen. Sappiamo che l'Unione europea, per quanto riguarda le materie prime critiche, dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, esponendosi così ai rischi elevati lungo la catena di approvvigionamento. Recentemente, com'è stato ricordato anche da altri colleghi, l'ISPRA ha aggiornato dettagliatamente le mappe di queste materie, mettendo in luce anche le potenzialità dell'Italia. Nel nostro sottosuolo, infatti, sono presenti almeno quindici delle trentaquattro materie prime critiche necessarie per la transizione energetica. Sono stati identificati circa 3.000 siti ed entro il 2025 è attesa la pubblicazione di una nuova carta mineraria aggiornata. È per questa ragione che il nostro Gruppo parlamentare al Senato, e prima alla Camera, ha cercato di migliorare il testo di questo decreto con emendamenti concreti, ponendo l'accento su temi come il riciclo dei rifiuti e degli scarti produttivi. Il problema di fondo, invece, è che questo provvedimento è mancante di coraggio e di visione, a cominciare dal fatto che ignora aspetti cruciali del regolamento europeo, come il riciclo dei rifiuti elettronici da cui potremmo invece recuperare risorse importanti per la nostra industria. Il comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche proposto dal decreto è eccessivamente concentrato su ricerca ed estrazione, senza misure adeguate sull'economia circolare. Preoccupa anche l'assenza nel decreto di norme chiare a proposito di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale; nemmeno si prevedono iniziative specifiche per l'approvvigionamento di materie critiche da riciclo. Insomma, a voler essere generosi, si potrebbe osservare che siamo di fronte ad un insieme di enunciazioni di principio incapaci di produrre effetti concreti. In realtà si fa ancora di peggio. Basti pensare che questo decreto-legge cancella il tavolo nazionale di lavoro per le materie prime critiche, che era operativo dal 2021, sostituendolo con una nuova struttura senza rappresentanti del mondo della ricerca, delle professioni specifiche e dell'industria. Insomma, lo fa mettendo in evidenza, ancora una volta, una scelta e un atteggiamento che vi è proprio e che riflette quella sindrome di occupazione del potere di cui questa maggioranza dà sistematicamente prova. Le disposizioni del decreto in esame sollevano interrogativi critici riguardo le competenze regionali e la partecipazione delle comunità locali nelle decisioni che influenzano direttamente i loro territori. riguardo, colleghi, voglio dirlo ancora una volta: da un lato, predicate l'autonomia differenziata assegnando tra le ipotetiche ventitré materie anche l'energia alle Regioni, scelta che io penso sia sbagliata e oggi fuori dal tempo; dall'altro lato, però, centralizzate i processi decisionali rischiando di creare un cortocircuito tra competenze statali e regionali, che evidenzia ancora una volta come la vostra sia inconsapevolezza o inadeguatezza o improvvisazione. *(Applausi)*. Scegliete voi. Non c'è però dubbio che vi dovete chiarire su questo punto: volete l'autonomia differenziata o la centralizzazione delle decisioni e delle competenze? Vi dovete chiarire al vostro interno, perché è evidente che ci sono spinte diverse se guardiamo i singoli provvedimenti. Di questo il Paese si accorge e il cortocircuito rischiate di crearlo davvero. Infine, per concludere questo mio intervento, voglio ricordare le parole di un grande europeista, Altiero Spinelli, commissario europeo all'industria che, durante la Conferenza di Venezia del 1972 (mi piace ricordare che quella conferenza si tenne proprio a Venezia), pose con ferma autorevolezza questa questione. Nel suo intervento era forte il richiamo all'atmosfera di insicurezza dovuta alla rilevante dipendenza europea in quasi tutte le materie prime. Sottolineava Altiero Spinelli l'inadeguato livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la posizione di forza dei fornitori che erano in grado di condizionarci, avvertendo in maniera davvero visionaria la minaccia nel lungo termine di una penuria delle materie prime. Ecco, oggi ci troviamo esattamente in quella situazione: le guerre e le tensioni geopolitiche hanno reso ineluttabile la realtà rispetto alla quale Spinelli ci aveva messo in guardia. queste vostre misure sono davvero insufficienti e non sono adeguate ad affrontare questa sfida. Andrebbe migliorata la conoscenza delle caratteristiche geologiche, stimolato il tessuto industriale, rafforzata la capacità diplomatica di ogni singolo Paese e del nostro. La ripresa delle attività di ricerca e di coltivazione mineraria dovrebbe avvenire come una vera e propria scelta industriale ma - come è stato detto - integrando ricerca, trasferimento tecnologico e formazione. Pertanto, ribadisco la nostra ferma critica e annuncio il voto contrario del Gruppo Partito Democratico rispetto a un provvedimento cercato di dire - pericolosamente contraddittorio, che non risolverà i problemi di un settore tanto decisivo per l'economia nazionale. Pur non potendo ormai più aspettarci molto da voi, sarebbe davvero quanto mai opportuno che la maggioranza considerasse seriamente i punti da noi sollevati e che lo facesse per il bene della nostra economia e del futuro industriale del nostro Paese.

siamo qui oggi per votare il decreto-legge sulle materie prime critiche di interesse strategico. Il decreto in esame affronta un tema di fondamentale importanza per il futuro del sistema produttivo nazionale. In particolare, introduce norme urgenti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento dell'Unione europea dello scorso aprile, mirato a garantire un adeguato sistema di approvvigionamento di metalli e minerali che, per la loro dislocazione geografica, per problemi nelle negoziazioni commerciali fra Paesi, nonché per la sussistenza in aree geografiche turbolente, non sono facilmente accessibili. L'Unione europea stima che nel 2030 l'Europa avrà bisogno diciotto volte in più di litio e cinque volte in più di cobalto rispetto ai consumi attuali, per la fabbricazione di batterie per veicoli elettrici e stoccaggi di energia. Come è noto, queste materie si trovano all'interno dei dispositivi elettronici che usiamo quotidianamente, ma sono anche alla base di tecnologie particolarmente innovative che agevolano le nostre vite, come fibre ottiche, laser, di molte apparecchiature che aiutano specialmente l'ambiente, per esempio con le batterie per le auto elettriche, i sensori elettrici, i convertitori catalitici indispensabili per la produzione di tecnologie *green*, come turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Queste materie prime critiche oggi sono per lo più estratte al di fuori dell'Unione europea. È reale il rischio che nei prossimi anni l'Europa potrebbe trovarsi impossibilitata nel raggiungimento di obiettivi relativi alla transizione ecologica e a quella digitale, tematiche che stiamo portando avanti anche grazie al lavoro del Governo rispetto al raggiungimento degli obiettivi legati alle misure del PNRR. Non si tratta di una posizione politica, poiché l'interesse nazionale dovrebbe essere interesse di tutti, in maniera trasversale. Quel che è certo è che lo è per il Governo di Giorgia Meloni. Continuiamo a vedere la Cina protagonista nella produzione di settori chiave della transizione energetica: solare, eolico, produzione di batterie con più dell'80 per cento della capacità mondiale. Pensate solo al fatto che la media delle tempistiche per ricevere l'autorizzazione per l'attività estrattiva in Europa è tra i nove e i dodici anni, mentre in Cina bastano soltanto tre mesi. Il sistema che istituisce questo decreto-legge agisce anche sulla rapidità e, quindi, permetterà di accorciare le distanze del principale *competitor* d'Europa. Questo decreto risponde bene al Regolamento europeo. Innanzitutto ci consente di recuperare una parte importante dell'industria italiana come quella mineraria, ferma da decenni. In questo periodo di tempo il mondo e altri Paesi europei si sono organizzati, mentre l'Italia ha visto i siti minerari diminuire drasticamente e non per esaurimento delle risorse, ma a causa delle convenienti condizioni dei mercati esteri e per la mancanza di lungimiranza della politica industriale mineraria del passato. passato. L'Italia non ha più soddisfatto il fabbisogno di materie prime critiche, ma ha prodotto perlopiù materiali utili all'industria del vetro, della ceramica, quando invece gli esperti minerari riuniti dal servizio geologico d'Italia ritengono che nel Paese esistono ancora diverse aree con ottime potenzialità minerarie anche in relazione alle materie prime critiche. L'Italia, inoltre, è all'avanguardia nell'industria del riciclaggio, che assume particolare importanza se si tiene conto che molte miniere chiuse o abbandonate dispongono ancora di materiale di risulta precedentemente non preso in considerazione, e che oggi, invece, vista la necessità di svincolarsi dall'estero e di aumentare l'indipendenza nazionale ed europea, è essenziale per recuperare da esso elementi ancora utilizzabili.

Si tratta di un decreto-legge che favorisce notevolmente l'attenzione in tema ambientale, particolarmente caro - se vogliamo - alla sinistra che pone un voto contrario, anche se in maggioranza europea. europea. Continuiamo allora a non capire quale sia il vostro impegno concreto su queste materie oltre all'ideologia. Sarebbe stato un gesto di grande responsabilità sociale, di buonsenso e di rispetto verso gli italiani se oggi aveste votato anche voi convintamente un'azione legislativa così efficace e innovativa. Non è così. A voi manca quel senso probabilmente di responsabilità politica che serve alla Nazione, come avete dimostrato in più occasioni e dimostrerete ancora oggi. Noi invece continuiamo orgogliosamente a lavorare affinché questa Nazione non resti spiazzata o inerte, come è accaduto in passato. Signor Presidente, fatte queste considerazioni, riteniamo che le materie prime critiche siano oggi il petrolio e il gas del futuro. Questo decreto-legge propone un nuovo approccio all'approvvigionamento, che sarà fondamentale per sviluppare la domanda e l'offerta del futuro e aiuterà l'Italia soprattutto a non Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Signor Presidente, il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione. Nel complesso, i dati di consuntivo mostrano nel 2023 un generale miglioramento dei saldi, sia rispetto alle previsioni iniziali sia rispetto alle previsioni definitive. Dalla gestione di competenza del 2023 si rileva, infatti, come si sia registrato un miglioramento dei saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio del 2022, ad eccezione del ricorso al mercato. In particolare, il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, presenta nel 2023 un valore negativo di circa 124,6 miliardi di euro, con un miglioramento di 5 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2022. Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali di circa 29,8 miliardi, pari a circa il 4,2 per cento, che ha compensato il lieve aumento delle spese finali di 24,8 miliardi, pari a circa il 3 Quanto al risparmio pubblico, che rappresenta il saldo delle operazioni correnti e che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale, esso si attesta nel 2023 a 42,9 miliardi di euro, con un miglioramento di oltre 17,1 miliardi rispetto al 2022. Infine, si fa presente che il dato del ricorso al mercato finanziario, che misura la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti, si attesta nell'anno 2023 a un valore negativo di circa 402,5 402,5 miliardi di euro, superiore di circa 11 miliardi rispetto al dato del 2022, ma inferiore di circa 109 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e di circa 132 miliardi rispetto alle previsioni definitive. Nel complesso, i risultati della gestione 2023 denotano per tutti i saldi un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive, anche considerando gli scostamenti autorizzati dal Parlamento in corso di esercizio. Essi risultano, inoltre, rispettosi dei limiti massimi autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023, come successivamente aggiornati. A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2023, che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali di circa il 4,2 pari a 29,8 miliardi di euro, rispetto all'anno precedente, accompagnato da un lieve aumento anche degli impegni e delle spese finali di circa il 2,9 per cento, pari a 24,8 miliardi di euro rispetto al 2022. Guardando alle operazioni complessive, comprensive delle entrate per accensione di prestiti delle spese per rimborso prestiti, la gestione di competenza 2023 denota un aumento degli accertamenti di entrata complessivi del 9,3 pari a 94,6 miliardi rispetto al 2022, e un aumento degli impegni complessivi di spesa del 3,7 per cento, pari a oltre 40,9 miliardi. Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio 2023 ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 741,6 miliardi di euro, con un incremento a consuntivo di 4,2 punti percentuali, pari a 29,8 miliardi rispetto al dato riferito al 2022. Gli accertamenti sono risultati superiori a quanto prospettato di circa il 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali, per le quali l'importo atteso era pari a 672,3 miliardi a 672,3 miliardi di euro e di circa il 9 per cento rispetto alle previsioni definitive, per le quali l'importo stimato era pari a circa 680 miliardi. L'incremento degli accertamenti di entrate finali è derivato interamente dall'aumento registrato dalle entrate tributarie, mentre le entrate extratributarie e le entrate per alienazione e ammortamento dei beni hanno fatto registrare una riduzione di accertamenti. Per quanto riguarda i dati di consuntivo relativi alle spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si fa presente che i relativi impegni nel 2023 si sono attestati a 866,1 miliardi di euro, registrando un incremento di circa circa 24,8 miliardi, pari al 2,9 per cento. Si segnala, a tal proposito, che all'interno di tale aggregato la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 695,3 miliardi di euro, in aumento di 14,2 miliardi rispetto al 2022; mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa 10,6 miliardi, attestandosi a 170,9 miliardi di impegni. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per circa 278 miliardi di euro, con un aumento del 6,17 per cento rispetto al dato del 2022, quando i rimborsi erano stati pari a 261,8 miliardi, gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.144 miliardi di euro, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente di circa il 3,7 per cento. Assumendo a riferimento i valori di previsione, si evidenzia come i dati risultanti dalla gestione siano risultati inferiori sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni per quanto riguarda tanto le spese finali, quanto le spese correnti, mentre le spese in conto capitale, stimate in 157,7 miliardi di euro nelle previsioni iniziali, sono risultate pari a 170,9 miliardi a consuntivo. Con riferimento alla gestione dei residui, si rivela che anche nel 2023 il loro ammontare continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate, sia dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella relazione al rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti e precedenti registrava al 1° gennaio 2023 residui attivi per un valore di 235.337 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per per 193.495 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 41.843 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate in misura pari a 89,31 miliardi di euro, sia dal lato delle uscite con una riduzione di 52,33 miliardi, di cui circa 5,3 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. Pertanto, il saldo attivo tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 era pari a 41.843 milioni di euro, per effetto delle variazioni intervenute nell'anno si è ridotto a 4.860 milioni, con una flessione di 36.982 milioni

Il rendiconto 2023 registra 105.280 milioni di euro di residui attivi di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2023, e 57.603 milioni di euro di nuovi residui passivi. Nel complesso, dunque, i residui attivi al 31 dicembre 2023 risultano pari a 251.306 milioni, mentre i residui passivi al 31 dicembre 2023 ammontano a 198.769 milioni. Nel complesso, quindi, il conto dei residui al 31 dicembre 2023 presenta una eccedenza attiva di 52.537 milioni di euro. Si ricorda che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Si segnala che, in termini di cassa, il saldo netto da finanziare è risultato pari, nel 2023, 173 miliardi di euro, con un incremento di 10,5 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente, in cui il saldo si era attestato a 162,5 miliardi. Si evidenzia come la gestione di cassa abbia complessivamente dato luogo, infatti, a incassi complessivi per per 1.050,1 miliardi e a pagamenti per 1.128,7 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2022, un aumento sia degli incassi, del 3,2 per cento, che dei pagamenti, del 2,3 per cento. In particolare, gli incassi finali evidenziano un aumento di 21,4 miliardi di euro rispetto al 2022, attestandosi a 679,1 miliardi, a fronte dei 657,7 registrati registrati l'anno precedente. Il volume dei pagamenti finali si attesta a 852,2 miliardi di euro, con un aumento di 31,9 miliardi di euro rispetto al 2022. Il conto generale del patrimonio, le cui risultanze sono riportate nell'articolo 6 del disegno di legge, comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità bilancio e quella patrimoniale. Si evidenzia altresì come dai risultati generali della gestione patrimoniale 2023 emerga un'eccedenza passiva di circa 2.758 miliardi, con un peggioramento di circa 163 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2022, pari in termini percentuali al 6,3 Il totale delle attività ammonta a circa 1.048,6 miliardi, con un aumento di 7,3 miliardi, mentre il totale delle passività ammonta a 3.806 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Nel segnalare che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2023, con l'esclusione da tale da tale dichiarazione di alcuni capitoli delle entrate e delle spese, si rinvia per maggiori approfondimenti al riguardo alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e del Senato. Da ultimo, si rileva come, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 36,

alla spesa primaria per i programmi ambientali ammontano a circa 25,8 miliardi, pari al 2,6 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Si registra quindi una riduzione della spesa ambientale rispetto al dato relativo al 2022, che tuttavia faceva riferimento anche alle misure per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale. Per ulteriori approfondimenti rimandiamo appunto al *dossier* n. 351/1 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

perché sono stati stressati, enfatizzati, sottolineati e volutamente resi protagonisti di questo assestamento. Innanzi tutto, vi è il miglioramento del saldo netto di 169 milioni, dato che fa capire quali siano la tenuta dei conti pubblici e il lavoro che il Ministero dell'economia e finanze sta svolgendo, per cui ringrazio il Governo, presente in Aula nella persona del sottosegretario Albano. l'aumento delle entrate (16,4 miliardi), per di più di natura tributaria. Il risparmio pubblico di quasi 18 miliardi (17,9, per la precisione) rimane certamente un saldo negativo, ma da 69,2 miliardi si arriva a 51,6. Variazioni importanti ne abbiamo avute durante l'anno.

nazionale e internazionale, i conti del bilancio di previsione, con un cambiamento che si è registrato per quanto riguarda i fondi per la Protezione civile, alla luce degli eventi alluvionali del 2023 che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche; un assestamento focalizzato sul realismo e sulla responsabilità, che va a verificare le effettive entrate e le effettive spese previste, adeguando i conti pubblici alle necessità e senza compromettere la stabilità finanziaria del Paese. L'efficienza della spesa pubblica è un altro tema tenuto in debita considerazione, frutto di un'analisi approfondita e puntuale delle priorità nazionali. Si va a investire laddove occorre e dove realmente è necessario; così sulle politiche di sviluppo. L'assestamento rispecchia la volontà di sostenere le politiche economiche e sociali, con un focus particolare sull'innovazione tecnologica, la transizione ecologica e la formazione professionale, e un'adeguata attenzione sulla trasparenza e sulla partecipazione. Sulla trasparenza vorrei fare qui i

arrivare a capire immediatamente quali sono le poste in campo e soprattutto qual è stato il lavoro messo in cantiere. E ciò anche per quanto riguarda il bilancio di previsione, che andremo a scrivere dall'autunno di quest'anno, soprattutto alla luce delle regole di contabilità, che sono state modificate e che potrebbero mettere in crisi un sistema che però, stando a questi conti e alla loro tenuta, non fa intravedere alcuna frattura. In conclusione, agli onorevoli colleghi dico che questo assestamento di bilancio - ve lo dice una persona che lo ha letto, lo ha verificato, lo ha consultato e lo ha studiato non è soltanto un atto formale, ma è anche un atto programmatico, che dà chiari segnali di tenuta dei conti pubblici. Pertanto, è un passo deciso per un futuro stabile ed equo per tutti i cittadini italiani. crescita economica e coesione sociale. Chiedo a tutti di fare una valutazione obiettiva e oggettiva su questo lavoro, valutando tutti, compresa la minoranza, la possibilità di votare favorevolmente.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale, con la presenza del numero legale, dei disegni di legge rendiconto 2023 e assestamento 2024 avranno luogo alla ripresa dei lavori. Sospendo la seduta fino

Questa mattina si è conclusa la votazione degli articoli del disegno di legge di Rendiconto. Poiché al disegno di legge di assestamento non sono stati presentati emendamenti ed esso si compone del solo articolo 1, passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul

perché in realtà, a parte il clima già un po' da pre-vacanza, non c'è molto da dire. Sicuramente non stiamo parlando di un provvedimento che lascerà il segno nella storia. a me sembra opportuno precisare una serie di considerazioni doverose nell'ambito di un'analisi politica un po' più generale. Noi stiamo andando avanti con questo Governo senza intervenire in modo strutturale sulle storture e sui problemi che il Paese ha e che condizionano un esercizio, in termini di politica di bilancio, che sia dirottato verso le esigenze prioritarie del Paese stesso. Quindi, meno si affrontano i nodi strutturali e meno sarà questo Governo in grado di intervenire nell'ambito delle politiche che davvero necessiterebbero al Paese: sanità e riforme di vario genere. C'è un dato che deve essere in qualche modo sottolineato. È il dato dell'aumento delle entrate tributarie. Anche qui è un bel mistero: si continua a dire che non ci sono interventi in termini fiscali, che non ci sono prelievi ulteriori, ma questi dati vanno considerati nell'ambito di una politica complessiva. Non si riesce a capire come il Governo riuscirà a garantire quei tagli, ad esempio i tagli sul cuneo, che dovranno essere confermati nella legge di bilancio. Continua ad aumentare la spesa pubblica, senza un minimo di riflessione su possibili *spending review* che potrebbero essere fatte, continuando a danzare sul Titanic come se non accadesse nulla o non ci fossero altre possibilità di intervento. Vi sono poi delle questioni particolarmente odiose, nell'ambito di una strategia più complessiva che riguarda il Paese e il suo sviluppo. Ad esempio, avete dimezzato le risorse sulla diversificazione delle fonti energetiche. Per un Governo che pone il tema energetico come centrale, questa è una notizia che deve essere necessariamente rilevata.

nella quale abbiamo evidenziato tutti i problemi infrastrutturali del Paese. Ad agosto, noi abbiamo un Paese in tilt, che non riesce a muoversi, con i turisti che ci guardano con occhi sgranati perché non siamo in grado di garantire neppure un servizio. Però, i tagli sui trasporti e sulle infrastrutture sono sempre una priorità assoluta per questo Governo, nel quale si sbraita molto, si litiga come maggioranza, si prova a fare gesti di forza in una direzione o nell'altra, ma un dato è chiaro: Salvini non tocca palla.

sul tumore al seno. Colleghe e colleghi, questo provvedimento prevede quasi un milione di tagli ai test genomici per il carcinoma mammario. Questa cosa non può passare inosservata, perché chi siede in Commissione bilancio si ricorderà la battaglia che in piena notte abbiamo fatto per avere un aumento dei test, che sono ovviamente funzionali al tema della prevenzione e della lotta a uno dei tumori più diffusi e anche più mortali.

E non mi si venga a dire che è perché non si riuscivano a spendere queste risorse, perché, se non si riesce a spendere su un tema così importante, il problema lo avete voi

a quello del debito), ma ci sono delle coordinate nei tagli che fanno capire qual è la priorità di questo Esecutivo. A maggior ragione, dal momento che che la questione della prevenzione del tumore al seno è, a mio modo di vedere, uno dei temi su cui noi dobbiamo impegnarci di più nei prossimi anni, chiedo ancora una volta, proprio per evitare che la politica dei tagli del Governo vada avanti, di sottoscrivere la mozione che abbiamo presentato e di rimettere al centro della discussione di quest'Aula una priorità assoluta per le donne e per tutti i cittadini.

Qualcuno potrà dire che non è una novità; certamente, anche perché questo rendiconto è in linea con il DEF che abbiamo contrastato abbiamo espresso un giudizio negativo, anzi, per alcuni versi, i segnali sono addirittura peggiori rispetto alla situazione. Voi date importanza, ad esempio, alla questione occupazionale; in termini di numeri avete ragione, purtroppo, in termini di ore lavorate, no. C'è qualcosa che non funziona; se aumenta l'occupazione, ma diminuiscono le ore lavorate, vuol dire che ci sono dei problemi molto seri

e i salari non hanno alcuno strumento, tranne alcuni pochi contratti, ed elementi di recupero della questione inflattiva. Dall'altra

se vogliamo guardare avanti, non possiamo continuare a dare il messaggio che i giovani devono continuare a vivere nell'instabilità permanente, fondata sulla deregolamentazione del proprio rapporto di lavoro e quindi sui *voucher* e sui contratti a termine,

Siete contro il salario minimo, non prevedete alcun elemento di recupero dal punto di vista della perdita inflattiva,

del viaggio fatto recentemente dal Presidente del Consiglio con un gruppo di industriali, ad esempio, ci viene detto

che vanno verso il 2 per cento. Se voi pensate che l'economia si possa rilanciare esclusivamente con l'aumento delle spese militari, esportando

La domanda è la seguente: le tasse devono continuare a pagarle solo lavoratori dipendenti e pensionati, o anche quelli che hanno guadagnato tanti soldi in questi anni?

a questo, ci sono imprenditori illuminati che non si scandalizzano se viene messa una piccola patrimoniale, perché in una situazione di difficoltà tutti dovrebbero andare in questa direzione. In tutto questo, oggettivamente non c'è non c'è alcuna inversione, quindi, in sostanza, come dicevo all'inizio, noi confermiamo il nostro voto contrario perché, anziché migliorare o ascoltare le cose che abbiamo detto quando abbiamo discusso del Documento di economia e finanza

che la gestione dei conti pubblici non solo è stata prudente, ma anche virtuosa, credo che anche i colleghi della minoranza dovrebbero farsene una ragione. Nel 2023 tutti i saldi sono migliorati sono migliorati sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto a quelle finali. Il prodotto interno lordo cresce di 123 miliardi di euro, passando dai 1.962 del 2022 ai 2.085 miliardi del 2023. In conseguenza della crescita del prodotto, tutti i dati del rendiconto misurati in rapporto al PIL sono migliori rispetto a quelli precedenti. Inoltre, ci sono circa 94,5 miliardi di entrate in più anno su anno tra il 2023 e il 2022, di fronte a un aumento di spesa di quasi 41 miliardi.

cosa per la quale si è lavorato, sia attraverso le imposte sostitutive sui redditi degli autonomi. Le spese quindi aumentano, ma crescono meno delle previsioni iniziali e anche questo evidenzia una gestione prudente dei conti pubblici. L'assestamento 2024 prevede maggiori entrate per 26,7 miliardi utilizzate per 19,5 miliardi per maggiori contributi agli investimenti. Inoltre, scende il valore della spesa pubblica rispetto al prodotto interno lordo; la destinazione delle nuove spese, anche dopo la rimodulazione delle voci di spesa esistenti, si sposta soprattutto verso il sostegno alle attività delle imprese italiane. L'Irpef in crescita, grazie ai redditi dei nuovi lavoratori, è il segnale che l'economia cresce aumentando il numero degli occupati, arrivato a un nuovo *record*. C'è una evidente crescita dell'economia dei servizi, che colma l'attesa della ripresa del settore industriale, i numeri dell'assestamento del primo semestre 2024 proiettati sull'intero anno consentono di ragionare con una maggiore possibilità di analisi persino sui numeri della manovra di bilancio. Purtroppo, la speculazione cerca e ha cercato di innescare anche notizie false su nuove tassazioni sui profitti delle banche, tasse che non ci saranno. Il nostro sistema produttivo ha bisogno del sostegno importante dei nostri istituti di credito che puntualmente daranno il proprio credito all'economia reale, avendo già rafforzato i propri requisiti patrimoniali. Il Governo esce quindi premiato dai due anni di Governo fotografati da rendiconto e assestamento. Sulla base di questi dati si intravede una manovra di bilancio che confermerà le misure in favore dei redditi medi e a sostegno del sistema Italia. due disegni di legge, il rendiconto 2023 e l'assestamento 2024, che contengono numeri sicuramente positivi e per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

abbiamo visto tutti la felicità della *premier* Meloni e di tutti i componenti del Governo e della maggioranza, ma ci siamo chiesti cosa c'è dietro questi festeggiamenti. Eppure è sotto gli occhi di tutti: la spesa sull'attuazione del PNRR è lenta, va a passo di lumaca.

Diamo per buono il dato fornito dal Ministro, ma 52,2 miliardi rispetto ai 102 miliardi di euro arrivati ed erogati dall'Unione europea a quanto Non lo dice Ketty Damante, lo dicono i numeri: sì e no siamo al 50 per cento della spesa effettuata sui 102 miliardi ottenuti. Eppure, dall'attuazione del PNRR dipende il 90 per cento della crescita di quest'anno, il 2024, almeno così ha scritto il Governo nel DEF, cui l'apporto positivo del piano al PIL, proprio quello di cui parlava il collega che mi ha preceduto, importantissimo, si mantiene vigoroso anche nel 2025, con l'83 per cento, e nel 2026, con il 73 quindi, abbiamo ottenuto 102 miliardi, ne abbiamo spesi soltanto 52 ed entro giugno 2026 - e siamo già ad agosto 2024 - ne dobbiamo spendere 143. 143. Credo che non sia sfuggito a nessuno dei presenti in quest'Aula, compresi i colleghi della maggioranza, che proprio ieri la *premier* Meloni, felice e contentissima, ha comunque legato il versamento della Commissione europea e l'incasso della rata proprio proprio all'ultimo dato sul PIL fornito dall'Istat, che ha registrato una crescita dello 0,7 per cento nel primo semestre del 2024. Se però non attuiamo la spesa, non spendiamo e rimangono i soldi nei cassetti, non ci sono né crescita e credo che questo Parlamento, oggi che discute rendiconto 2023 e assestamento 2024, una riflessione la debba fare. *(Applausi)*. Non c'è nulla da festeggiare, siamo tutti molto preoccupati.

un periodo di tempo infinito per una delle economie più sviluppate del mondo e per un sistema Paese come l'Italia, che non ha mai conosciuto un periodo così lungo di contrazione

attribuiva alle politiche economiche dal Governo Conte il disastro e il crollo della produzione industriale di allora. Se il Governo oggi però dispone di questi scienziati, me la faccio una domanda: ma com'è che non hanno nemmeno pensato a impostare uno straccio di politica economica quegli scienziati che trasudavano astio a ogni parola nelle loro accuse a una politica economica errata, ma che almeno c'era? Adesso che sono al Governo è forse lo stesso amor di patria di prima che impedisce loro di vedere diciassette mesi di regressione industriale. Colleghi, crescita e PNRR hanno un unico denominatore, l'impatto sulla legge di bilancio, ma anche la tenuta dei conti pubblici, perché la mancata attuazione del PNRR potrebbe compromettere e aumentare i ritardi della spesa, e quindi le erogazioni future. Questo ce lo dice l'Unione europea, non lo dicono

il Governo intensificherà il monitoraggio sull'attuazione. Io l'ho percepito quel messaggio realistico e lo dovremmo percepire tutti quanti noi qui in Parlamento che non è tutto oro ciò che luccica e che è soltanto propaganda di facciata dire che tutto va bene in Italia. In meno di due anni dobbiamo portare a casa tutti gli obiettivi

che portano a ritardi e l'amministrazione centrale. Il Ministero delle infrastrutture è fermo al 15 per cento e che diciamo delle erogazioni ai Comuni? Ecco perché noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo fatto una proposta di legge, l'istituzione di una Commissione di vigilanza, perché ha ragione il ministro Fitto: dobbiamo intervenire di più sulla vigilanza e sul controllo dell'attuazione, perché non si scherza più. Tra l'altro, ci sono troppe incertezze. Il ministro Fitto parla di revisioni al PNRR. Ancora revisioni? Ancora revisioni? O, ancora, il ministro Giorgetti parla di chiedere una proroga. Il PNRR va portato a casa, ora o Ecco che vi stiamo dando una mano con l'istituzione di questa Commissione di vigilanza e controllo. Ma basta dire che siamo i primi, Non basta dire che siamo i primi e voglio dire con onestà che noi siamo i primi ad aver ottenuto cinque rate, ma non diciamo - almeno il Governo non lo dice che noi siamo quelli che abbiamo avuto più soldi e quindi abbiamo più rate da incassare. Altri hanno avuto di meno, ma sono più veloci, vedi la Francia. vedi la Francia. In alcuni rapporti, ad esempio il rapporto percentuale tra scadenze già raggiunte e il totale di quelle previste, al primo posto c'è la Francia, lo sapete dov'è l'Italia? Al nono ma il Governo non lo dice ed esulta per le erogazioni, che è tutt'altra cosa che l'attuazione. E potrei continuare all'infinito, ma l'unica cosa che rimane certa e su questo io credo, colleghi, dobbiamo fare una riflessione, opposizione e maggioranza - è che la leva sulla crescita è al momento spuntata.

Io non so quali atti avete letto; io ho letto il *dossier*, anche se in Commissione non è che ne abbiamo discusso poi così tanto. Il quadro generale degli andamenti dei saldi di competenza in valore assoluto mostra un generale peggioramento delle previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali, con dati allarmanti, legati essenzialmente ad un sostanziale aumento delle previsioni di spesa di circa 24,8 miliardi di euro, a cui fa riscontro un lieve aumento delle corrispondenti previsioni di entrate (28,8 miliardi). Ma c'è un debito pubblico aumentato di 170 miliardi di euro. Poi, quanto all'assestamento, la volontà del Governo è sempre orientata nel senso di rinviare al prossimo mese di settembre l'adozione delle principali scelte di fondo di politica economica. Si aspetta il piano strutturale di bilancio di medio periodo, da presentare entro il 20 settembre. Ecco, Presidente, queste motivazioni, ma soprattutto la mancanza di attenzione alla crescita della produzione industriale e all'attuazione del PNRR, non possono che farci votare contro questo provvedimento.

mi rendo conto che rendiconto e assestamento non sono esattamente degli argomenti che scaldano i cuori, specialmente in questo periodo dell'anno. Effettivamente concordo, sono due documenti tecnici su cui il Parlamento può intervenire poco, perché si tratta più che altro di prese d'atto di situazioni contabili.

contingente. Sapete com'è la nostra vita, ma forse il nostro lavoro si conosce poco all'esterno: siamo sempre di corsa, presi per questo o quel comma da approvare in una Commissione, la Commissione di merito, il parere e così via. Passiamo poco tempo, secondo me, a riflettere assieme su quale potrebbe essere un'idea differente dell'economia o della gestione di uno Stato. Questa idea differente dovrebbe essere da parte nostra, in quanto Parlamento, trasmissibile al Governo. Non vorrei sinceramente che quest'Aula - e parlo anche per la maggioranza - tenda a un atteggiamento che a me non piace, che è quello della passività nei confronti dell'andamento del Governo. Noi dovremmo essere propositivi e per essere propositivi ognuno di noi, che ovviamente ha contatto diretto e indiretto con i nostri colleghi che in questo momento sono al Governo, dovrebbe essere, secondo me, conscio di quello che si può fare. Quello che si può fare ci viene detto dai numeri del rendiconto e dell'assestamento, perché se prendiamo i numeri del rendiconto, vale a dire dire l'esito finale dei conti del 2023, guardando quell'esito, senza esagerare senza esagerare con i dettagli, penso che ci sia una cosa che salta all'occhio a tutti, vale a dire cos'erano le previsioni e cos'è l'attualità. Le previsioni davano molto banalmente un *deficit* molto più basso

- questo per i motivi che ben sappiamo, superbonus, soprattutto, comunque spese maggiori rispetto al preventivato - e il rapporto debito-PIL è andato al 137

elemento è la crescita in questo caso, in un tessuto arido come quello di tutti gli Stati europei, ma soprattutto dell'Italia, che non ha investimenti, che non ha spesa da tempo,

sicuramente avremmo potuto fare infrastrutture, centrali, energia e interventi di questo tipo e avremmo ottenuto esattamente lo stesso meccanismo di crescita del PIL, ma anche più duraturo.

gran voce che l'Italia ha bisogno di investimenti e noi dovremmo insistere per riuscire ad averne sempre di più rispetto ad ora, perché il nostro arretrato in termini di investimenti è così alto che ogni goccia in più che viene versata dà frutto e dà segni positivi. Cosa abbiamo invece nell'assestamento? L'assestamento ci indica un valore che salta all'occhio ed è stato richiamato da tanti colleghi, che in questo caso ci insegna come dobbiamo fare: ci sono 16,4 miliardi in più di entrate tributarie,

Direi proprio di no, perché le tasse - tutti lo sanno - non le abbiamo aumentate. Da dove arrivano i 16 miliardi in più? Derivano da un miglioramento delle condizioni economiche e soprattutto dal fatto che magari tanta gente non è più nel reddito di cittadinanza, ma è nel lavoro vero Guarda caso, l'aumento si è registrato soprattutto nell'Irpef. Da dove arriva l'Irpef, secondo voi? Ovviamente arriva dal fatto che c'è un numero maggiore di occupati. Questo numero maggiore di occupati dà come risultato un gettito fiscale più alto e quindi

raggiungeremmo sicuramente non con più tasse ma con più crescita, e questi dati ce lo stanno dimostrando. Si cresce anche senza avere un aumento fortissimo del PIL, ma semplicemente sistemando qualche stortura che c'era nel passato, come nel caso del passaggio da un'economia di sussidio

Quando la gente sarà molto contenta di andare a sanare delle vecchie e piccole irregolarità all'interno del proprio appartamento pagando una determinata cifra, ecco che si avrà questa curiosa magia della gente che paga volentieri le tasse, perché in una maniera o nell'altra le cose migliorano. migliorano. Questo è un obiettivo che si può ottenere. Penso che stiamo facendo un buon lavoro e che questi dati ci testimoniano come bisogna fare e qual è la strada da perseguire. Noi contiamo di andare avanti su questo binario, perché i numeri ci stanno dando ragione. la discussione del rendiconto e dell'assestamento rischia di essere un passaggio un po' burocratico. Cerco di prendere spunti dai numeri per fare il punto su alcuni nodi di politica economica in una fase peraltro delicata: l'Italia è in procedura per *deficit* eccessivo; la Commissione europea ha trasmesso al nostro Paese la traiettoria di riferimento che sarà la base per costruire il piano strutturale di bilancio che va consegnato entro fine settembre. Anzi, Presidente, colgo l'occasione per nuovamente al Governo che venga resa pubblica la traiettoria comunicata dalla Commissione europea, per mettere tutti in condizione di fare le proprie valutazioni. In questa fase è utile, credo, fare qualche riflessione su questi nodi di politica economica. Il primo riguarda le entrate fiscali, a un anno dall'approvazione della legge delega. La riforma è stata varata con grandi ambizioni e il vice ministro Leo ha fatto persino riferimento alla riforma Cosciani del 1972-1973. A un anno di distanza e dopo parecchi decreti attuativi, possiamo dire che quello che è venuto fuori è molto lontano da quelle ambizioni e soprattutto molto lontano da ciò che servirebbe al Paese. I mali del nostro sistema fiscale li conosciamo, ma di fronte ad essi la riforma, stando a quello che abbiamo visto, ha prodotto risultati molto modesti. L'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef ha prodotto otto euro di tasse in meno al mese, peraltro solo per il 2024 e vedremo se questo intervento proseguirà; la tanto sbandierata deduzione aggiuntiva Ires per un anno e invece l'abolizione permanente dell'ACE, dell'aiuto alla crescita economica, che comporterà un aggravio strutturale di quasi tre miliardi di euro di tasse in più per le imprese. Invito tutti a leggere un recente rapporto Istat: la deduzione Ires beneficia poco più del 5 per cento delle imprese. L'abolizione ACE aumenta le tasse per oltre un'impresa su quattro in questo Paese. Non è esattamente un intervento per rafforzare la competitività del sistema produttivo. *(Applausi)*. Signor Presidente, stendiamo un velo pietoso sulla lotta all'evasione fiscale, sull'innalzamento al tetto dei contanti, sulle sanatorie e i condoni, sulle rottamazioni, le proroghe delle rottamazioni, fino alla pantomima del redditometro e - mi si conceda l'espressione - ai saldi di fine stagione sul concordato preventivo biennale, con la pia illusione - come ha detto qualche giorno fa la mia collega Tajani - di fare cassa, di chiedere qualche soldo in più ai contribuenti interessati, ma continuando a strizzare l'occhio a una parte del proprio elettorato. Le due cose non stanno insieme e, nonostante gli ammorbidimenti progressivi, lo strumento non è destinato ad avere un grande successo. Insomma, sul versante fiscale quella che è stata fatta è una riforma fallimentare, prigioniera della vostra propaganda e del blocco sociale che la destra vuole continuare a difendere. Questa difesa a oltranza, però, avrà come unico risultato quello di rendere ancora più ingiusto e inefficiente il nostro sistema fiscale; aggraverà la debolezza dell'economia italiana e non permetterà a voi di trovare le risorse che servono per finanziare servizi essenziali a partire dalla sanità, che è in una condizione di drammatica sofferenza. secondo punto, signor Presidente, riguarda l'attuazione del PNRR. Ieri è arrivata la quinta *tranche*, di undici miliardi di euro, salutata, come sempre, da un entusiastico commento della Presidente del Consiglio. Questa retorica trionfalistica è scollegata dalla realtà e, soprattutto, è scollegata da quanto il ministro Fitto ha raccontato al Parlamento pochi giorni prima, quando ha ammesso che, su 194 miliardi del Piano, finora, a meno di due anni dalla scadenza, ne sono stati spesi 52: 52 miliardi su 194, con la messa a terra dei progetti in forte ritardo e con dati sconfortanti sulle missioni inclusione e coesione e salute. Sottolineo quest'ultimo punto sulla salute, con la messa a terra del 10 per cento delle risorse attribuite: un doppio danno per la sanità pubblica, perché mancano fondi per la parte corrente e tutte le Regioni sono in sofferenza. Dove sono i soldi per gli investimenti, per fare gli ospedali, per comprare i macchinari, per migliorare la sanità pubblica? Questi soldi messi a disposizione dal PNRR non li state spendendo e stiamo sprecando un'occasione d'oro per dare una sanità migliore agli italiani. Vogliamo parlare del piano Transizione 5.0? Lo avete annunciato nove mesi fa e siamo a zero. Non un euro è stato erogato alle imprese per sostenere i loro investimenti, perché il decreto attuativo è stato firmato solo venerdì dal Ministro per il Made in Italy e queste risorse, che sarebbero preziose per sostenere le nostre imprese, non sono ancora state utilizzate: alla faccia dei proclami di politica industriale. in poco meno di due anni noi dovremmo spendere 140 miliardi di euro, avendone spesi solo 52 a fine luglio del 2024. Non sarebbe più utile, signor Presidente, concentrarci su questo punto, anziché commentare entusiasticamente l'arrivo della quinta rata? È una domanda retorica, ma è una sollecitazione forte che noi vogliamo rivolgere al Governo. Il terzo punto concerne la spesa pubblica. Ho ascoltato il ministro Giorgetti all'assemblea dell'ABI. il Ministro ha sottolineato, come spesso fa, la volontà del Governo di realizzare una seria politica di controllo della dinamica della spesa pubblica.

di chi riceveva il reddito di cittadinanza. Avete lasciato a piedi 700.000 famiglie di questo Paese. *(Applausi)*. Il secondo esempio riguarda il lavoro del Mezzogiorno. Noi avevamo introdotto la decontribuzione Sud e voi state ponendo termine a quella misura, certo risparmiando. "Risparmierete" oltre 14 miliardi di euro nei prossimi otto anni, ma lo fate facendo cassa sulle imprese e sui lavoratori del Mezzogiorno. Il terzo esempio concerne le pensioni. Altro che riforma delle pensioni! La deindicizzazione che avete fatto con la legge di bilancio per il 2023 vi fa risparmiare quest'anno 4 miliardi e 100 milioni e, nei prossimi otto anni, 30 miliardi e 600 milioni di euro. Voi state facendo cassa sui pensionati *(Applausi)* e la vostra revisione della spesa è a danno dei poveri, dei lavoratori del Mezzogiorno, delle imprese e di chi sta in pensione. ultimo punto, avviandomi alla conclusione, sulla vicenda di questi giorni: le dimissioni del Ragioniere generale dello Stato. Dobbiamo parlare anche di questo passaggio dopo mesi di polemiche e di pressioni. È stato citato il superbonus negli interventi di tanti colleghi. Presidente, in un Paese normale spetterebbe alle forze politiche, economiche e sociali fare autocritica per quello che è successo. Tutte le forze politiche hanno votato le proroghe e l'estensione di quella misura. In Italia no: è stato individuato un capro espiatorio che è stato poi sacrificato. Detto questo, si pone un tema molto delicato che riguarda i criteri e le procedure per l'individuazione del nuovo Ragioniere generale. Non è una questione da poco. Per ricoprire questo incarico non serve un fedelissimo del Ministro di turno: serve una figura caratterizzata dalla massima autorevolezza e dalla massima indipendenza *(Applausi)*. Parliamo infatti di una funzione chiave per la verifica dei conti pubblici. Per questa ragione chiediamo nuove regole. Le consuetudini del passato non bastano più. Avete occupato militarmente tutte le postazioni di responsabilità, volete occupare anche questa, servono nuove regole a tutela del Paese. In conclusione, Presidente, siamo in una fase nuova. A fine settembre il Governo dovrà presentare il piano strutturale di bilancio. Dovrebbe essere quella l'occasione per indicare la rotta dei prossimi sette anni. Visto quello che è successo in questo anno e mezzo, abbiamo di che essere molto preoccupati. Avete messo in campo una politica economica rinunciataria; avete fatto una riforma fiscale corporativa e iniqua; non avete fatto le politiche industriali che servirebbero per rilanciare la crescita, facendo cassa sul sociale, sulle pensioni e sui lavoratori. I numeri del Rendiconto e dell'assestamento certificano queste scelte sbagliate. Ed è sulla base di questi motivi che annuncio il voto contrario del Partito Democratico sul Rendiconto generale

della riforma della *governance* europea che effettivamente - ricordo - nessuno dei partiti ha votato, perché indubbiamente la traiettoria che prima il senatore Misiani ci chiedeva di vedere insieme sarà molto complicata e difficile da rispettare. Del resto, addirittura la Corte dei conti ieri ha chiarito che ci sarà una grande difficoltà, per esempio, nel mantenere quella che è la spesa in ambito sanitario a causa della traiettoria che ci viene chiesta da Bruxelles

Il parere è stato favorevole, per esempio, rispetto alla grande preoccupazione che evidentemente da quei magistrati veniva rappresentata sulla voce economica della sanità, che invece noi abbiamo voluto mantenere ai livelli più alti di sempre, nonostante i profeti di sventura parlassero di un calo della spesa in ambito sanitario.

il dato che ci viene fornito dagli Uffici e che noi ci stiamo accingendo a votare è positivo: l'incidenza degli stanziamenti complessivi sul PIL è diminuita di sei decimi nel complesso; il saldo netto da finanziare, data la differenza fra le entrate fiscali e le spese finali, nel 2023 presenta un valore negativo di 124 miliardi, con un miglioramento, però, di 5 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2022. E tale miglioramento è frutto - devo dire che mi ha fatto piacere sentirlo dalle parole pronunciate dai senatori dell'opposizione - anche dell'extragettito straordinario che vi è stato grazie a delle riforme che hanno reso il fisco

stabilità. Procedendo nella disamina di questi dati molto rilevanti, noi crediamo che uno degli elementi relativi all'economia reale su cui avevamo l'esigenza di intervenire

secondo cui vi è stato un incremento eccezionale del lavoro in Italia. E vi è stato perché il Governo Meloni non ha fatto altro che applicare una ricetta semplice,

sostituita con un sostegno alle categorie veramente vulnerabili e svantaggiate della società, andando invece a riportare i nostri giovani al centro, a lavorare insieme alle donne e a tutti coloro che stanno partecipando partecipando alla rimessa in piedi dei conti italiani. *(Applausi)*. Purtroppo, noi non riusciamo ad accettare lezioni a livello di politica economica da chi

che avevamo studiato e ipotizzato in precedenza e che stiamo raggiungendo, nonostante le notevolissime difficoltà.

impresa. Ma forse ciò deriva dal fatto che vi sono difficoltà nelle catene produttive e, siccome il Governo lo sa bene, ha scelto di andare ad incrementare del 6,6 per cento gli impegni rispetto al passato esercizio, prevalentemente imputabile ai maggiori impegni per categorie dei contributi agli investimenti alle imprese. Qualche altro senatore, prima, si preoccupava del fatto che non vi fosse una ricaduta sulle amministrazioni comunali e locali degli impegni delle nostre manovre di bilancio. Ma vorrei tranquillizzarli ricordando loro che abbiamo avuto un incremento dell'1,2 per cento rispetto al dato del 2022 dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche locali e previdenziali. Ricordo che a un mio primo intervento circa due anni fa fui felice di annunciare che a Roma, per esempio, la Capitale d'Italia, abbiamo fatto arrivare 2,3 milioni euro per la realizzazione di un'infrastruttura finanziata all'epoca con una legge obiettivo che non ha mai visto la luce con i sindaci del MoVimento 5 Stelle e purtroppo ancora con i sindaci del PD. E allora, quando qualcuno di voi rappresenta preoccupazione perché i fondi non vengono utilizzati in modo adeguato, lo pregherei di portare la sua preoccupazione - sicuramente sarà meglio ascoltato da lui di quanto non sia ascoltata io - al sindaco del PD, già Ministro dell'economia, Gualtieri della nostra Capitale d'Italia. La città oggi è in una condizione di cantierizzazione

insorge. Vorrei concludere dicendo che siamo lieti e felici di consegnare il voto favorevole di Fratelli d'Italia al Rendiconto e all'assestamento di bilancio e di continuare a essere vagoni di testa a livello economico europeo.

Senatrici, senatori, tra due giorni - le nostre sedute

Faccio riferimento a quella maledetta mattina del 1956, quando nelle miniere di carbone belghe scoppiò un incendio che causò 262 vittime; di quei minatori morti, 136 erano nostri compatrioti, erano italiani, figli della nostra Italia, andati lì in cerca di fortuna, in cerca di lavoro più che di fortuna, in cerca di un reddito con un lavoro molto duro, che potesse garantire il sostentamento delle loro famiglie perlopiù rimaste a casa, in Italia. Erano italiani prevalentemente del Centro e del Sud, ma erano figli della nostra comunità nazionale. È per tale motivo che questa tragedia è diventata simbolo del coraggio della resilienza e della forza di volontà di un popolo disposto a compiere qualsiasi rinuncia perché animato da un forte desiderio di riscatto sociale e di mettersi di mettersi duramente alla prova col lavoro per garantire un futuro ai propri figli. Noi quel momento fondante della nostra comunità - perché è tale - lo ricordiamo

non l'abbiamo mai dimenticato, nemmeno le istituzioni lo hanno mai dimenticato. Anche il nostro Presidente della Repubblica ha avuto modo negli anni passati di ricordarlo. E mi mi consentirete un ricordo personale, relativo a un ex ministro della Repubblica parlamentare,

anni, ad essa vogliamo rifarci. Se Tremaglia si inginocchiava, anche noi oggi, simbolicamente, ci inginocchiano davanti a quei caduti del lavoro, che esprimono la volontà ancora oggi esistente nel popolo italiano di andare avanti anche con il sacrificio dei più umili. A loro dedichiamo qualche attimo di silenzio.

di quelli che non ci sono più e hanno lasciato le loro anime, la loro esistenza, i loro sogni, le loro speranze e le loro famiglie in fondo a quelle gallerie.

c'erano tanti abruzzesi, molisani e anche veneti. Ricordo personalmente da bambino che, quando tornavo in Cadore dalla famiglia di mio papà, ce n'erano tanti che tornavano dal Belgio ed erano quelli che venivano in Italia nelle loro case e raccontavano di quel buco e di quel botto, ma anche di come a quei tempi nei bar e negli esercizi pubblici ogni tanto si trovasse la scritta «Vietato l'ingresso ai cani e agli italiani». Vedete,

che ha vissuto sofferenze immani: siamo stati un popolo di emigrati, ma che ha sempre rispettato, ha dato e ha voluto dare. Mi inchino a quelle vittime e ricordo tante cose: ricordo di esserci stato tante volte con Tremaglia, che volle far sì che l'8 agosto fosse celebrato ogni anno come il giorno del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. …lo dobbiamo proprio a quell'intuizione e a quella volontà, che è un fatto di riconoscenza, ma anche di orgoglio e di bellezza, nonostante tutto, nel dolore, ricordando gli italiani che hanno combattuto di più per fare comunque grande la nostra Patria.

stasera prendo la parola per ricordare il sessantottesimo anniversario del disastro minerario di Marcinelle, la più grande tragedia mineraria a colpire la nostra emigrazione in Europa. Come lei stesso ha detto, Presidente, la mattina dell'8 agosto del 1956, nella miniera del Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, un incendio causò la morte di 262 persone, di cui 136 immigrati italiani. Il disastro minerario di Marcinelle fu il terzo più grave in termini di vittime italiane, dopo quelli di Monongah e di Dawson negli Stati Uniti, con un bilancio pesantissimo per tutta la comunità italiana. Ancora oggi le nostre comunità nel mondo portano il peso di queste tragedie, per sempre scolpite nella nostra memoria. Noi siamo gli eredi di quelle vicende, della sofferenza di chi ci ha preceduto, di chi ha sacrificato la propria vita per dare un futuro migliore alla generazione successiva. Abbiamo dunque il dovere di onorare la memoria delle vittime e di non disperdere il valore del loro sacrificio, soprattutto per i nostri giovani, così che anche loro conoscano un pezzo importante della nostra storia e apprezzino i privilegi di cui godono oggi. Perciò l'8 agosto, giornata dedicata al sacrificio del lavoro italiano nel mondo - ma non soltanto l'8 agosto credo che abbiamo il dovere di unirci, come Paese, in un pensiero di gratitudine per tutti i nostri connazionali che furono costretti a lasciare il proprio Paese, la propria famiglia e tutto ciò che per loro era sicuro e familiare per lo sconosciuto, rischiando tutto per la speranza di un futuro migliore. Il mio auspicio, Presidente, per l'8 agosto dell'anno prossimo e per tutti gli 8 agosto a seguire, è che questa storia venga raccontata non soltanto dagli italiani nel mondo, ma anche dagli italiani in Patria, per dare il giusto riconoscimento a chi ha dato un tributo alto, spesso la vita stessa, al miglioramento della propria Patria in momenti difficili e allo sviluppo dei Paesi di accoglimento. Facciamo tutti in modo che il sacrificio del del lavoro degli italiani nel mondo non sia avvenuto invano e che la nostra gratitudine si traduca in impegno per il futuro. Signor Presidente, voglio unirmi anch'io al ricordo di quei connazionali e della loro tragica fine, ricordando che il momento in cui persero la vita in quella miniera era il culmine di una sofferenza e di un dolore, del fatto di essere stati costretti a lasciare le loro case e di dover arrivare in un Paese straniero, di cui non conoscevano la lingua. Erano persone che lavoravano in situazioni intollerabili, senza sicurezza - come è stato già detto - e che persero la vita proprio perché le condizioni di lavoro in cui si trovavano erano disumane. Dobbiamo ricordare - io credo - il lavoro italiano nel mondo utilizzando questa importante data nazionale, ma estendendo l'omaggio a i tantissimi nostri connazionali che sono emigrati nei cinque continenti. Non dobbiamo mai dimenticare che tanti italiani lasciarono tutto il Paese, e non soltanto il Sud, ma anche tante Regioni del Nord, per andare in Sudamerica, in Europa, in Australia, per andare davvero dappertutto. Io penso che questo ci dia una responsabilità ulteriore: guardare con rispetto a tutte quelle popolazioni e a tutte quelle persone che oggi

italiani avevano da sopportare. Spero che questa giornata di riflessione non passi invano e ci ricordi che siamo stati un Paese di emigranti e abbiamo avuto opportunità da altri Paesi. che il nostro occhio nazionale guardi oggi a coloro che cercano un futuro qui da noi, come avremmo voluto che gli altri Paesi che ci ospitarono guardassero ai nostri migranti di quell'epoca.

delle 136 vittime. Mi piace ricordare - come diceva nella parte iniziale il collega Scalfarotto - i tanti emigranti che hanno portato il valore dell'Italia nel mondo. Se la

Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia mi associo alle sue parole, che meglio di ogni altro intervento hanno espresso un cordoglio generale e un ricordo alle vittime di Marcinelle, ma anche al richiamo che lei ha fatto all'impegno per la sicurezza sul lavoro oggi, che quelle vittime ci spingono ad assicurare. Non dobbiamo darci tregua fino a quando oggi, in Italia e nel mondo, la sicurezza sul lavoro non sarà garantita a tutti. Con questo spirito ci uniamo alle sue parole e rendiamo omaggio alle vittime di ieri, nell'auspicio che non ce ne siano mai più domani in nessuna parte del mondo. *(Applausi)*.

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 i senatori Bazoli, Berrino, Boccia, Borghi Borghi Claudio, De Cristofaro, Liris, Lisei, Malan, Paita, Patuanelli, Romeo, Ronzulli, Spagnolli, Zaffini e Zullo.

di Servigliano, nelle Marche. Quel campo oggi è monumento nazionale grazie ad una legge di cui ho l'orgoglio di essere primo firmatario. Robert tenne un diario dal novembre del 1941 al settembre del 1944, che racconta la sua cattura, la prigionia nel campo di Servigliano, l'evasione, l'arrivo in Piemonte,

Questo diario, a cui Robert volle dare un titolo evocativo, «Servigliano Calling», è a tutti gli effetti un documento storico unico ed eccezionale: racconta la vita del campo, la durezza estrema, ma anche i sogni e le speranze, i momenti di socialità come le partite di calcio, e raccoglie le poesie e i disegni dei compagni di prigionia di Robert.

Presidente. Leggere quelle pagine ha grande significato, per capire ed avere consapevolezza dell'enormità di una storia che è la nostra storia fondativa, che ci riguarda e ci appartiene. Quel diario è stato ritrovato, custodito per decenni, prima da una giovane ragazza piemontese innamorata di Robert e poi dai familiari di Robert, e da loro è stato consegnato alla "Casa della memoria" di Servigliano. Intorno a quel diario, le scuole del territorio stanno portando avanti progetti didattici. C'è un lavoro sulla memoria che rinsalda il legame con le nuove generazioni e che va implementato in ogni scuola, in ogni Comune, perché sempre si sappia da quale lotta gigantesca - e a quale costo sovrumano - derivano la democrazia e la libertà che oggi abbiamo. Robert, lasciati i campi di prigionia, restò in Italia e fece la sua scelta di vita: si unì ai partigiani che combattevano il fascismo, perché gli ideali di democrazia, di eguaglianza e di libertà sono universali e non hanno confini. Robert è stato trucidato il 5 marzo 1945, a pochi giorni dalla liberazione. A Robert Dickinson e ai partigiani di ogni sentimento (comunisti, socialisti, cattolici, liberali, azionisti) che seppero trovare la forza morale di essere antifascisti noi dobbiamo tutto ciò che siamo, noi dobbiamo la nostra Repubblica. A loro noi dobbiamo la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza. *(Applausi)*. *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è inammissibile come questo Governo, con il decreto-legge *tax credit*, stia distruggendo la piccola impresa, quella impresa caratteristica dell'imprenditoria italiana, spesso di tipo familiare, che ha costituito il fiore all'occhiello delle aziende del *boom* economico. Mi riferisco in particolare ai settori dell'intrattenimento audiovisivo e dei grandi eventi culturali. Non è un caso che, a seguito dell'approvazione del decreto *tax credit* audiovisivo, lo scorso 10 luglio tutti i lavoratori della filiera, e cioè le *troupe*, gli autori, gli attori i registi, abbiano animato una dura protesta contro un provvedimento scellerato. Mi chiedo: ma si è fatto quanto disse il presidente Giorgia Meloni in un noto discorso in Sicilia, a Catania, il 26 maggio 2023, quando affermò la lotta all'evasione non si fa al piccolo commerciante, dal quale vuoi il pizzo di Stato? In quel contesto, inoltre, affermò anche che non avrebbe disturbato chi ha voglia di fare. Bisogna prendere atto che non solo non si è fatto ciò che il presidente Giorgia Meloni ha detto, ma si è attuato tutto il contrario. Signor Presidente, attraverso lei, mi rivolgo alla Presidente del Consiglio. Io auspico che la *Premier* dedichi un maggiore impegno a questa categoria. Sono certa che la presidente Giorgia Meloni, che precedentemente ha distrutto la Via della Seta, piuttosto che cimentarsi nel commentare costantemente episodi di cronaca - come nel caso degli incontri di *boxe* femminile tra Angela Carini ed Imane Khelif - farà ciò per cui è stata eletta, ovvero tutelare gli interessi di tutti gli italiani. Reputo sacrosanta l'azione di denuncia dei numerosi sindacati, testate e siti di settore, tra cui Cometa Rossa. Di fatto, il Governo ha cancellato il *tax credit* per le piccole e medie imprese.

È necessario che il Governo si attivi per istituire un tavolo di confronto con tutte le associazioni di filiera. Anzi, auspico che il ministro Sangiuliano, con la sua sensibilità, possa anche farsi promotore di un dialogo costante con un settore che, da decenni, sta valorizzando a livello planetario la nostra industria audiovisiva. Mi riferisco al settore dei festival cinematografici. Onorevoli colleghi, poiché il tempo è tiranno, mi limiterò a ricordare il festival di Giffoni Valle Piana. Ricordo che nel 1982, l'indimenticabile regista François Truffaut, ospite

alle migliaia di ragazzi e ragazze che annualmente popolano questo evento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cultura non ha e non dovrà mai avere un colore politico. La cultura è patrimonio dell'umanità e ogni tentativo di scalfirla mina le fondamenta su cui si reggono le future generazioni.

io voglio in qualche modo richiamare l'attenzione verso un fatto molto grave, avvenuto pochi giorni fa, il 29 luglio, con missiva di minacce di morte inviata al pubblico ministero Luca Tescaroli:

Lo Stato deve dire no, deve esprimere solidarietà a quest'uomo della giustizia, a quest'uomo che combatte la mafia, che rischia la vita; e un uomo che, in un attimo di solitudine, pur avendo la scorta da tanti anni - una vita che, comunque, non augurerei a nessuno si chiude nella propria abitazione e magari pensa che sta lavorando per i cittadini, sta lavorando per l'Italia, sta lavorando per la libertà e la sua vita è a disposizione di tutti. tutti. Dobbiamo dire grazie a quest'uomo e dobbiamo esprimergli solidarietà. Io, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, la esprimo a pieno titolo al pubblico ministero, al dottor Tescaroli, all'uomo Tescaroli. Grazie! Grazie! Diciamo no alla malavita, no alla mafia, no a chi vuole uccidere colui che cerca la giustizia per tutti noi.